finestra"). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il nuovo calendario dei lavori per le prossime due settimane, fino a giovedì 12 febbraio. Per questa settimana restano confermati gli argomenti già previsti. Oggi pomeriggio inizierà la discussione del decreto-legge recante misure urgenti in funzione anticrisi, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi al fine di assicurare la votazione finale entro la seduta antimeridiana di mercoledì 28 gennaio, data di scadenza del provvedimento. Sono stati ripartiti inoltre i tempi per la discussione della relazione sullo stato della giustizia, già prevista nella seduta pomeridiana di mercoledì 28, che potrà proseguire oltre il consueto orario di chiusura. Le proposte di risoluzione dovranno essere presentate entro la fine della discussione generale. Nella seduta antimeridiana di giovedì 29 gennaio sarà esaminata la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella circoscrizione Estero. La prossima settimana si aprirà, martedì 3 febbraio alle ore 11, con la discussione del disegno di legge di ratifica del Trattato di amicizia Italia-Libia per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 29 gennaio. Seguirà l'esame della ratifica della Convenzione ONU sulla disabilità. Riprenderà quindi la trattazione, sospesa il 15 gennaio scorso, degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica. In tale occasione la Presidenza chiederà al Ministro dell'interno - come sollecitato da diversi Gruppi di intervenie sui recenti avvenimenti che hanno riguardato il centro di identificazione ed espulsione di Lampedusa connessi anche al tema degli sbarchi clandestini. Si passerà poi all'esame dei due decreti-legge, presentati in prima lettura al Senato, rispettivamente in materia di proroga termini legislativi e in materia ambientale, per i quali i tempi sono stati contingentati. La discussione di tali provvedimenti potrà proseguire nella settimana successiva, dal 10 al 12 febbraio, nel corso della quale saranno esaminati anche i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Per quanto riguarda la ripartizione dei tempi tra i Gruppi sui vari provvedimenti compresi nel calendario, la Presidenza favorirà una distribuzione non strettamente proporzionale, alla luce delle richieste avanzate dai Gruppi di opposizione, attraverso cessioni da parte di altri Gruppi. Il calendario sarà integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni. Nella seduta pomeridiana di giovedì 12 febbraio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

finestra") *(PD)*. Signor Presidente, in questi giorni stiamo assistendo, increduli e impotenti, ad un crescendo di episodi di violenza contro le donne iniziato oggi, ma che oggi è ancora più intollerabile: aggredite, stuprate, intimorite dalla violenza che le circonda e che è sempre in agguato quando rincasano, quando sono sole o no. Esse sentono la propria vita minacciata nella sua libertà e nel suo diritto elementare alla sicurezza. È un'emergenza vera per l'Italia; è uno scacco - duole dirlo - per il Governo, perché evidentemente non basta l'esercito nelle città, si tratti di 3.000 o di 30.000 uomini. Altre politiche sono necessarie affinché cresca nella società il rispetto verso le donne e verso la loro dignità. però ancora più increduli di fronte al commento di ieri del Presidente del Consiglio, il quale aggiunge verbalmente violenza a violenza: quella del linguaggio, appunto, della parola, che fa ironia sull'angoscia e sul dolore delle donne e per questo li rende insignificanti. infatti, ha radici nel costume e nella cultura ed è lì che essa deve essere combattuta, non alimentata. dire che ci vorrebbe un soldato per ogni bella ragazza italiana tradisce una cultura arcaica, reazionaria, secondo la quale lo spazio pubblico e la sicurezza di una donna non esistono in se stessi, non esistono se la donna non è accompagnata da un maschio. La coscienza di sé, del posto degli uomini e delle donne nella società, delle loro relazioni, La coscienza di sé, del posto degli uomini e delle donne nella società, delle loro relazioni, è uno dei temi della costruzione di una nuova Italia civile, moderna, gentile. Questo attiene al profilo di civiltà dell'Italia contro il suo imbarbarimento: possibile che non ci stia a cuore questa Italia? Il Presidente del Consiglio deve essere all'altezza di questa domanda e di questo compito. Siamo sgomenti, perciò, di fronte all'insostenibile leggerezza del nostro *Premier*, perché egli ci rappresenta di fronte al mondo. Davvero non ci interessano le battute; forse ad un po' di maschi sì, può darsi, ma alle donne sicuramente no. C'è proprio poco di cui sorridere nell'Italia di oggi e certamente non c'è niente Occorre soltanto consapevolezza, determinazione ed amorevole cura per le ferite dell'Italia, tra cui quella di cui stiamo parlando. Signor Presidente, chiediamo al Governo che ci venga a dire con serietà e responsabilità che cosa intende fare per contrastare l'aggressione in atto alle donne del nostro Paese. Dovremmo aprire, signor Presidente, una speciale sessione di lavori parlamentari per condurre in porto, con urgenza, leggi che attendono da anni - come quelle contro le violenze sessuali e le molestie diffuse nella vita pubblica e privata o, ancora, quelle per e finalmente politiche che valorizzino la capacità di lavoro delle donne e ne sostengano maternità e servizi sociali. È un intero orizzonte culturale e sociale, oltre che penale, che deve essere sostenuto, solo dal Parlamento e dal Governo, ma anche dalla cultura, dall'informazione, dai *mass media* e da un grande piano di educazione, perché si comincia dall'infanzia a contrastare questi fenomeni. Una grande politica, dunque, e non una battuta occasionale.

tema debba farci riflettere e guardare da un'altra prospettiva innanzitutto al problema drammatico e specifico dello stupro e della violenza sulle donne, anche con riferimento all'accelerazione dei tempi di approvazione delle nuove norme che riguardano le molestie persistenti. sulla circostanza che questo tema è connesso alla sicurezza individuale e collettiva, che non può più essere oggetto di slogan e di strumentalizzazioni di questa o quella parte politica. Nella passata legislatura ha sbagliato chi su questi temi, anche con riguardo particolare ai fatti che sono accaduti a Roma, ha strumentalizzato per fini elettorali episodi gravissimi di violenza omicida; sbaglia chi oggi ripete questo tipo di atteggiamento. Signor Presidente, non è questa l'occasione adatta, ma mi sembra giusto rilevare che il tema della sicurezza deve essere sottratto allo scontro politico, perché riguarda lo Stato di diritto e in materia di diritti costituzionalmente garantiti il confronto fra le diverse parti politiche è obbligatorio,

In questa logica, signor Presidente, è chiaro che fanno sorridere e fanno amarezza le battute, perché, al di là della buona o malafede che non è qui in discussione, su alcuni temi, per quanto possano venire semplici e spontanee, non fanno proprio ridere. ridere. È chiaro infatti che ad una bella ragazza non si può dire che il suo modello di riferimento deve essere sposare un uomo ricco e magari farsi scortare da un militare dell'esercito. A mio avviso, oggi, anche per quanto riguarda le battute, le donne e gli uomini di questo Paese meritano qualcosa di più e

che inneggia alla violenza di gruppo, allo stupro e a quei signori, a quei mascalzoni, a quei farabutti che praticano questo tipo di violenza sulle donne. Come vede, è un tema che, purtroppo, torna di attualità (è di questa mattina l'ulteriore polemica con Facebook, per la verità non solo da parte mia, ma di tanti esponenti,

del peggio della cultura di distruzione della civiltà che esiste nel nostro Paese. Non è tollerabile, signor Presidente, non solo che continuino a esistere esistere gruppi a sostegno di Riina, di Provenzano o delle Brigate rosse, ma che a questi si siano associati gruppi a sostegno di coloro i quali operano stupri individuali e collettivi. Credo che tutto ciò ci debba ulteriormente far riflettere e la prego, signor Presidente, conoscendo e apprezzando la sua sensibilità di carattere istituzionale, di provocare anche nel Governo quel tanto di indignazione che basta ad assumere un'iniziativa non solo di controllo formale e rassicurante nei confronti di questi siti e di questi *social network.* Tuttavia, poiché credo che nel nostro Paese siamo in presenza di soggetti che sfuggono alle regole del diritto italiano

Credo sia giunto il momento in cui non soltanto il Senato, traendo spunto dal suo intervento, segnali la delicatezza di questa tematica al Governo (e le assicuro che lo farà immediatamente),

continuo a ribadire che stiamo discutendo di temi - credetemi - estremamente delicati. Adesso, il presidente D'Alia ne ha introdotto un altro, di pari delicatezza - e non mi permetto di dire più delicato di quello delicatissimo posto dalla senatrice Soliani

È un episodio sul quale credo che la politica, le istituzioni e il Parlamento siano chiamati a pronunciarsi, per fare in modo che si possano evitare questi scenari. Stiamo discutendo di questo, colleghi. Dicevo, presidente D'Alia, che la presenza del ministro Alfano nel dibattito che ci impegnerà nel pomeriggio di mercoledì potrà costituire un momento di riflessione,

dell'introduzione, all'interno di questi siti internazionali, di espressioni di posizioni estremamente pericolose, non solo per i nostri figli, ma anche per la quiete sociale. Signor Presidente, mi associo alle parole così trattenute che la collega Soliani ha trovato

Sulla natura dei fatti, credo si potrebbe aggiungere, a quanto la collega Soliani ha detto, la lettura dell'intervista dolente che Franca Rame ha rilasciato oggi al giornalista Fabrizio Roncone del «Corriere della Sera», quale riesce a trattare un argomento che ha conosciuto di persona con tatto e anche con una certa sapienza, quella della distanza. È istruttivo leggerla, perché da una voce che potrebbe inneggiare alla vendetta esce, invece, una parola di riflessione e di saggezza. Questo chiama in causa il saltare dei nervi che spesso si verifica di fronte a vicende di questo genere. Infatti, appena accade un fatto di questo tipo, viene fuori subito il meccanismo del

che deve riguardare la certezza della pena per chi compie questi atti, insinuando nell'opinione pubblica il fatto che già con la carcerazione preventiva si potrebbe determinare una punizione, mentre sappiamo che da questo punto di vista c'è un profondo errore giuridico. L'idea del farsi giustizia da sé poi innesca delle reazioni vaste, totalmente dislocate, come il caso in cui ignoti assalitori, facendosi forti di una violenza di gruppo esecrabile, sono andati a punire non perché quelli non li ha trovati nessuno, ma ha individuato un gruppo di rumeni come potenziali correi virtuali; c'è stata una sorta di assalto con una certa vocazione al linciaggio che dice troppe cose sul modo con cui la mentalità collettiva non sa trattenersi di fronte a fatti di questo tipo. L'esigenza di giustizia è una cosa, l'esigenza di linciaggio è completamente un'altra. C'è una sorta di pervertimento dei sensi dentro questo modo di affrontare gli argomenti e non aiuta la tecnica che appare abbastanza dominante nella gestione degli strumenti dell'opinione pubblica. Non voglio farne una tragedia, ma non posso fare a meno di ricordare che, nei mesi precedenti alle elezioni, il centrodestra, con i suoi mezzi di comunicazione e con la sua ampia disponibilità su questo terreno,

via - proprio a fini di competizione sulla scena elettorale. Il centrosinistra veniva fotografato come un Governo imbelle, che non riusciva a fronteggiare simili situazioni e si prometteva ovviamente un atteggiamento diverso da parte del centrodestra. Purtroppo si vede che, di fronte a fatti del genere, anche il centrodestra è totalmente impari, perché sono fatti che è difficile prevenire, è difficile controllare. In proposito, secondo me, non fa tanto scandalo la battuta infelicissima del Presidente del Consiglio che rivela più che altro una dimensione di subcultura; preoccupa piuttosto il fatto che i suoi mezzi di comunicazione, da decenni, abbiano rappresentato la donna, la femmina, la femmina bella, desiderabile, assaltabile, come un oggetto non oscuro del desiderio collettivo; questa idea che la donna, proiettata nella mente dell'uomo, del maschio aggressore, continuamente presente su tutte le pagine, su tutti gli schermi, in tutte le manifestazioni, in tutte le rappresentazioni... Voi avete un Presidente del Consiglio che è il proprietario di mezzi di comunicazione che da decenni... Può non piacervi, ma è la dura, schifosissima realtà. Avete un Presidente del Consiglio che possiede dei mezzi di comunicazione che, da decenni, esercitano un'influenza di pervertimento sull'opinione pubblica,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo preparato un intervento, ma mi riservo di farlo la settimana prossima quando affronteremo la discussione del disegno di legge sulla sicurezza.

per Roma e dintorni, ancora teatro di violenze. Dopo lo stupro della quarantunenne nella periferica zona di Primavalle, la scorsa settimana si è registrata l'aggressione di una coppia di fidanzati nelle campagne di Guidonia, alle porte della capitale,

Credo sia invece arrivato il momento che il Parlamento prenda delle decisioni e legiferi per bloccare o, perlomeno, limitare questi reati che si perpetuano costantemente ai danni delle donne. Credo anche non sia stato

Non voglio poi aggiungere tutto quello che si consuma tra le mura domestiche. Credo che oggi, presidente Schifani, non si possano

per rendersi conto che si tratta di un fenomeno che, anziché diminuire, continua, giorno dopo giorno, a crescere e questo non fa piacere. Penso non faccia piacere alle donne, ma neanche agli uomini, ai nostri compagni, ai nostri mariti o fidanzati.

il rispetto della dignità umana, della dignità della persona, costituisce il bene primario di ogni democrazia e di ogni azione politica, ogni misura volta a garantirlo e a tutelarlo deve essere da tutti sostenuta attraverso la cultura, attraverso la legge, attraverso la solidarietà. Il fenomeno della violenza sulle donne, che piuttosto che addolcirsi continua invece, purtroppo, ad inasprirsi, si può contrastare e combattere solo combinando contemporaneamente più azioni, tra cui, prima di tutto, l'attuazione di una vera e propria rivoluzione culturale, una presa di coscienza collettiva della società, che deve poi trasformarsi, come stiamo tentando di fare, in una battaglia comune di uomini e donne contro questa grave realtà. Sussidiarietà può essere una delle parole chiave: sussidiarietà tra Stato, ente locale, agenzie educative, associazioni e volontariato, così come si sta tentando di fare con le azioni del nostro Governo. A questo fenomeno deve poi aggiungersi un intervento sul piano legislativo, un intervento che è già in atto con la discussione sulla complessiva proposta contro la violenza sessuale del ministro Carfagna, perché alla gravità di questo fenomeno si si può davvero rispondere soltanto con un provvedimento articolato che non si limiti solo a sanzionare penalmente le molestie sessuali, ma sia sia soprattutto in grado di tutelare le donne contro ogni forma di violenza, favorendo la prevenzione, ma garantendo al contempo processi rapidi, accertamento della responsabilità e conseguente pena certa e adeguata per i colpevoli. Il reato di violenza sessuale - concordiamo pienamente con il ministro Alfano - è un reato gravissimo e altamente lesivo della dignità della persona, nonché della salute morale di chi lo subisce, e come tale deve essere giudicato. Questo è ciò che il Governo sta facendo grazie ai provvedimenti Bisogna poi lavorare sempre di più per dare alle donne la consapevolezza del loro diritto alla sicurezza e per intensificare la politica del sostegno alla vittima, perché una donna lasciata sola dalla società è una donna che subisce una doppia violenza. quindi tutte le colleghe, in maniera trasversale, a lavorare insieme tralasciando contrapposizioni sterili e limitando inutili polemiche per concentrarci sulle questioni vere per le quali servono proposte, fatti e azioni concrete. Il disegno di legge del ministro Carfagna prevede misure che rafforzano la tutela penale contro la violenza sessuale, introducendo aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole (ed è proprio questo di cui si sta parlando), imponendo l'aumento della pena in caso di recidiva e introducendo meccanismi volti ad accelerare i tempi di giudizio e la certezza della pena. provvedimento contiene norme volte a rafforzare la tutela contro la violenza sessuale tra le circostanze aggravanti, comportanti, per esempio, la reclusione da 6 a 12 anni; inoltre vengono ricompresi l'uso di sostanze comunque idonee a ridurre la capacità di determinarsi della vittima la qualità di ascendente e quant'altro. Il delitto di violenza sessuale e quello di violenza sessuale di gruppo vengono inseriti tra quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con le relative conseguenze sulla possibilità di celebrare il processo con il rito direttissimo ed immediato.

presa di coscienza di un fenomeno aberrante, come la volontà di alleggerire l'atmosfera in un momento di così grande tensione, come la volontà seria di intervenire. Non sono le battute a far male alle donne: è il silenzio, è la politica del non fare. Ribadisco: personalmente non mi sento offesa, senatore Pardi, ma mi sento stimolata ancora di più a combattere per il diritto alla sicurezza di tutte le donne, insieme alle colleghe, per prima Maria Ida Germontani, con la quale, da quasi vent'anni, combatto le le stesse battaglie all'interno del dipartimento delle pari opportunità del nostro partito.

oltre a quelle che sono state già introdotte nel cosiddetto disegno di legge sicurezza sulla violenza di gruppo, oltre a quelle che sono state già introdotte con il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati in materia di atti persecutori. Penso che una valutazione di esecrabilità

La violenza sulle donne va combattuta espressamente e principalmente sulla base culturale, educando le generazioni ad un nuovo tipo di rapporto, ad un nuovo rispetto della dignità della persona. Se su questo aspetto c'è la volontà del Parlamento, credo si possa trovare una soluzione in termini di sanzioni penali (se è necessario o meno, se è sufficiente o meno l'arresto domiciliare, che è pur sempre una misura cautelare preventiva).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, le previsioni economiche più recenti sono, come è noto ai più, particolarmente preoccupanti. Nell'area dell'euro, la frenata della domanda estera e la crisi dei mercati finanziari si sono innanzitutto ripercosse sulle decisioni di investimento delle imprese. Il clima di fiducia presso le imprese e le famiglie è ai minimi storici. Si diffondono i timori di un forte deterioramento del mercato del lavoro nell'anno appena iniziato. I principali analisti privati stimano in media un calo del prodotto di oltre l'1 per cento per il 2009. La Banca centrale europea, dopo la riduzione concertata di ottobre, ha ulteriormente abbassato i propri tassi di riferimento, nelle riunioni di inizio novembre e inizio dicembre, di 50 e 75 punti base, rispettivamente. Le aspettative di inflazione a breve e a medio termine, peggiorate in estate di pari passo con l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, si sono drasticamente ridimensionate negli ultimi mesi. Anche l'Italia è in recessione; le medesime previsioni scontano infatti una riduzione del PIL nel 2009 del 2 per cento e una ripresa solo nel 2010 con una crescita dello 0,5 Sono queste le previsioni della Banca d'Italia. Previsioni di un ulteriore peggioramento della crisi per il prossimo anno sono state avanzate anche dal Fondo monetario internazionale. L'occupazione, in crescita da oltre dieci anni, ha subito una battuta d'arresto nel terzo trimestre dell'anno scorso; si è intensificato nello scorcio del 2008 il ricorso alla cassa integrazione guadagni. A sua volta, il credito bancario cresce a tassi ancora sostenuti ma è in rallentamento, riflettendo una domanda di finanziamenti da parte di imprese e famiglie resa più prudente dalla recessione. Il rallentamento del credito è più intenso nei confronti delle piccole imprese. Sul fronte della finanza pubblica, gli effetti sui conti pubblici del peggioramento del quadro congiunturale sono inevitabilmente destinati a manifestarsi più fortemente nell'anno in corso, con un deficit che è previsto attestarsi al 3,8 per La manovra di bilancio per gli anni 2009-2011, di cui al decreto-legge n. 112, è stata integrata, senza modifiche significative, ai saldi programmati, con la legge finanziaria per il 2009 e con il decreto-legge in esame. Il decreto in esame reperisce risorse per 5,6 miliardi nel 2009 e le impiega essenzialmente per sostenere le famiglie con redditi bassi, per ridurre il prelievo fiscale sulle imprese e per stimolare l'attività di investimento. In relazione ai profili d'impatto sui conti pubblici, guardando alla composizione della manovra, l'effetto migliorativo dei saldi è essenzialmente riconducibile ad un aumento netto delle spese (principalmente di natura corrente) inferiore all'aumento netto delle entrate. Dal lato delle entrate, infatti, il testo in esame evidenzia un aumento netto decrescente tra il 2009 e il 2011. Le maggiori entrate derivano principalmente dalla rivalutazione dei valori contabili, complesso di misure che viene stimato comportare maggiori entrate significative nel primo anno di applicazione, nonché minori entrate per gli esercizi 2010 e 2011, dalle misure antievasione e per il recupero crediti delle amministrazioni pubbliche, dall'addizionale sul materiale pornografico e dall'aumento dell'IVA sui servizi televisivi. Relativamente alle minori entrate, è da segnalare l'introduzione della deducibilità dell'IRAP, le già citate misure di rivalutazione dei valori contabili, la detassazione dei premi di produttività e la previsione del pagamento dell'IVA alla riscossione del corrispettivo.

mentre le maggiori spese sono invece riconducibili al *bonus* per le famiglie (2.400 milioni di euro per il 2009), alle risorse a favore del trasporto ferroviario (480 milioni per ciascun esercizio del triennio di parte corrente, nonché 240 e 720 milioni per il 2010 e 2011 per gli interventi di parte capitale), all'integrazione del fondo occupazione (destinato a finanziare gli ammortizzatori sociali) e della legge obiettivo. In particolare, le misure contenute mirano, anzitutto, a contrastare le difficoltà economiche che, soprattutto, le famiglie e le imprese italiane incontrano in questa fase di acuta crisi economica, che, se di sicuro non ne pregiudica le prospettive di mantenimento, a medio termine, del benessere economico e sociale ad oggi raggiunto, le pone di fronte alle antiche e nuove carenze rispetto al modello di una moderna economia competitiva. In relazione al primo tipo di misure indicate in precedenza, va anzitutto segnalato il *bonus* famiglie, per cui si prevede che i cittadini residenti che compongono un nucleo familiare a basso reddito da lavoro dipendente o pensione o redditi assimilati riceveranno un *bonus* straordinario tra i 200 e i 1.000 euro, parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare e a seconda che in famiglia vi siano portatori di handicap*.* Inoltre, va segnalato il blocco delle tariffe per tutte le forniture abituali (fuorché l'acqua) fino al 31 dicembre 2009; per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le famiglie economicamente svantaggiate che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica avranno anche diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Di analogo tenore le misure volte al blocco dei pedaggi in aiuto ai lavoratori pendolari (sono bloccati i pedaggi autostradali e le tariffe ferroviarie sulle tratte regionali), nonché la concessione di un prestito (a tasso particolarmente agevolato) per le famiglie nel cui ambito avvengano nuove nascite, al fine di supportare le spese connesse alle esigenze dei primi anni di vita del nascituro. D'altro canto, nella linea delle azioni tese invece a rafforzare la tenuta patrimoniale dei nuclei familiari, va annoverata la previsione di un tetto agli oneri dei mutui per l'acquisto della prima casa, che non potranno superare il 4 per cento, e, per i mutui già stipulati, la previsione che lo Stato si accollerà l'eventuale parte eccedente. Sul versante delle imprese e dell'apparato produttivo in genere, vanno anzitutto considerate le riduzioni di tre punti percentuali dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la completa detassazione degli straordinari, con innalzamento da 30.000 a 35.000 euro del reddito massimo per beneficiare dell'aliquota agevolata e con innalzamento da 3.000 a 6.000 euro del salario di produttività agevolato fiscalmente. Inoltre, viene introdotto il sostegno in deroga al reddito di coloro che perdono il lavoro (cassa integrazione), le cui risorse saranno garantite dal nuovo Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nel quale confluisce anche il Fondo di occupazione per gli ammortizzatori in deroga, finanziato per 1.026 milioni di euro. Vi è poi la previsione per cui l'IVA verrà pagata d'ora innanzi dalle imprese al momento dell'effettiva riscossione dei corrispettivi. Vengono inoltre ridotti i costi amministrativi sostenuti dalle imprese e viene prevista la revisione degli studi di settore, soprattutto in talune aree del Paese, per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura. Al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, viene previsto che siano fiscalmente imponibili solo per il 10 per cento. Ulteriori interventi sono infine previsti a sostegno dei trasporti pubblici locali e delle ferrovie, insieme ad ulteriori misure di lotta e contrasto all'evasione fiscale che completano la manovra di sostegno all'economia. La strategia adottata dal Governo è stata, pertanto, quella di operare su due linee di intervento, dedicate, principalmente, a famiglie ed imprese, ma optando, nella selezione degli interventi prescelti, ad un approccio articolato in due fasi, affiancando, cioè, ad azioni aventi un impatto immediato (*social card*, *bonus* fiscale), interventi, invece, più generalmente rivolti al sostegno degli investimenti pubblici e privati nell'economia (cassa depositi e prestiti, sostegno ai mutui immobiliari) e all'innalzamento della produttività dei fattori. In tal modo, con il decreto in esame, si intende fornire un sostegno immediato alla domanda dell'economia, tramite, in particolare, le misure in favore delle famiglie, non tralasciando però azioni tese a potenziare e irrobustire i fattori da cui dipendono la tenuta ed il superamento della fase di crisi in atto: la competitività nei costi delle imprese e la produttività del lavoro. Nel suo complesso, sotto il profilo dell'impatto delle misure in termini di politica economica, lungi dall'esaurire l'ambito degli interventi in teoria necessari a fronte della gravità della crisi, la manovra lascia aperto il problema della quantità delle risorse che sarebbero indispensabili, innanzi tutto in termini di restituzione fiscale strutturale ai lavoratori ed ai pensionati, per un rilancio dell'economia sul versante di una vigorosa ripresa dei consumi. A tale proposito rammento che è già in corso una consultazione con le parti sociali sulle ulteriori misure da intraprendere nell'immediato futuro. È da segnalare, non di meno, che la manovra appare indubbiamente positiva come un primo intervento anticrisi a favore delle famiglie di pensionati e di lavoratori, soprattutto monoreddito e numerose, in maggiore difficoltà, per il miglioramento del salario dei lavoratori (anche quelli pubblici del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, con la detassazione consistente della parte collegata alla produttività), per la estensione degli ammortizzatori sociali a categorie che ne sono prive (compresi gli atipici) e, in ogni caso, per l'incremento dei relativi stanziamenti e per il sostegno delle imprese. Tutto ciò viene fatto preservando i saldi di finanza pubblica ed in attesa comunque di concordare eventuali ulteriori azioni in sede comunitaria, atteso che la congiuntura, come le più recenti previsioni confermano, avrà sensibili ripercussioni anche sul rispetto degli obiettivi programmati per il 2009.

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di cui oggi inizia in Aula la discussione per la conversione in legge, in legge, interviene sulla situazione di particolare crisi economica e finanziaria internazionale che ha colpito inevitabilmente anche il nostro Paese. È uno dei numerosi interventi in materia di risanamento della finanza pubblica, di agevolazione alla competitività delle imprese e di aiuto alle famiglie, che in questa legislatura hanno avuto avvio con l'approvazione del decreto-legge n. 112 del 2008, la cosiddetta manovra estiva, che pianificava in tre anni interventi per 36 miliardi di euro, per arrivare all'ottenimento del pareggio di bilancio entro il 2011, cioè entro il corso di questa legislatura, con la previsione, quindi, che già nel corso di essa il saldo primario di bilancio dello Stato possa consentire un'inversione di tendenza nella continua crescita del debito pubblico. Tali interventi sono poi proseguiti con l'approvazione della legge finanziaria e dei collegati che, voglio ricordare, hanno riguardato l'energia nucleare, il processo civile, la sburocratizzazione dello macchina dello Stato, gli interventi a garanzia della capacità di sostenere il credito da parte del sistema bancario. Questo è, viceversa, un intervento che riteniamo aggiuntivo a fronte di una manifestata capacità del Governo nazionale di anticipare molte delle risposte che la crisi internazionale richiedeva e che probabilmente in altri Paesi comunitari sono state assunte in ritardo rispetto alla formulazione tanto del decreto-legge n. 112 del 2008 quanto della manovra finanziaria dello Stato, il cui obiettivo di mettere in sicurezza la stabilità dei conti pubblici, per le dimensioni dell'indebitamento dello Stato italiano, assume carattere di evidente priorità. Onorevole Presidente, a beneficio dei colleghi e dell'efficacia del dibattito, preferisco consegnare agli atti una relazione che illustra nel dettaglio il provvedimento la cui discussione in quest'Aula inizia oggi. Desidero, infatti, cogliere questa occasione per svolgere alcune pur sintetiche considerazioni che, in qualche misura, diano conto del lavoro compiuto o, meglio, degli schemi di ragionamento che si sono snodati congiuntamente nelle Commissioni bilancio e finanze in queste settimane e delle riflessioni che, pare a me, ad essi possano conseguire. Desidero dare atto, innanzitutto, all'intera opposizione, che in Commissione ha cercato di andare al di là di una sterile contrapposizione. All'ordine del giorno abbiamo la conversione legge di un decreto che reca la data 29 novembre 2008. Va dato atto al Governo di aver previsto in tempo ciò che stava accadendo nei mercati internazionali. Le misure, il cui esame inizia oggi, vanno nella giusta direzione e credo sarebbe un errore pensare di poterle snaturare. Signor Presidente, colleghi, in questa Aula è avvenuto pochi giorni fa un fatto di straordinaria importanza: una riforma fondamentale, quella del federalismo fiscale, è stata approvata con pochissimi voti contrari. Per una volta maggioranza e opposizione non si sono prestate al gioco delle divisioni spesso artificiose. Bene, credo che quello spirito non vada disperso e che, anzi, a maggior ragione sia necessario oggi che iniziamo a discutere del sostegno che possiamo offrire alle famiglie e alle imprese del nostro Paese. Se riteniamo che questo provvedimento è - come è - un provvedimento giusto, non possiamo però negare a noi stessi che porta come data di origine il 2008. Sono passati solo due mesi, è vero, ma è come se fosse trascorsa un'eternità. La crisi infatti avanza e non aspetta i tempi del Parlamento. Convertire rapidamente questo decreto-legge e approfittare di questo dibattito per immaginare i prossimi passi è - credo - nell'interesse generale. Onorevoli colleghi, non possiamo ignorare che in queste ore si sta giustamente discutendo, nel Governo e nel Paese, delle nuove misure da intraprendere. Le imprese, ed alcuni settori in modo particolare, reclamano a gran voce un sostegno pubblico. Altri attori sociali chiedono di intervenire sul fronte dei consumi. Il Governo deve, a sua volta, garantire l'equilibrio dei conti pubblici. A nessuno può sfuggire che il nostro debito pubblico ci tiene con le mani legate. Certamente si potrebbe e si dovrebbe sfidare il tabù della spesa pubblica improduttiva e trovare lì le risorse che servono. Siamo in grado di violare interessi e incrostazioni consolidati? E ancora, ai colleghi dell'opposizione, che invocano un piano più massiccio di interventi pubblici, mi permetto di dire: troviamo insieme le coperture, mettendo al bando demagogia e populismo. Il presidente americano Barack Obama, così amato da tutti, ama ripetere che questa è l'era della responsabilità. È vero e tanto più lo è da noi. Responsabilità vuol dire che ci si muove in un sentiero stretto e che non disporremo di un'infinita quantità di denaro pubblico. Quindi, dovremo spendere al meglio quanto Governo e Parlamento riusciranno a mettere in campo. Dobbiamo essere attenti a non sprecare neanche un euro. Dobbiamo legiferare senza troppo forzare la mano invisibile del mercato ed avendo allo stesso tempo la piena consapevolezza che l'intervento pubblico serve solo se ha effetti moltiplicatori. Da questo punto di vista, dobbiamo sapere che la strada è obbligata ed è quella che ci consiglia di investire massicciamente in infrastrutture e in energia, in quella *green economy* che non corrisponde al vetero-ambientalismo andato di moda negli ultimi anni in Italia e in Europa. Mi riferisco alla possibilità di fare investimenti che offrano dividendi ambientali, ma anche economici. Affermare che il futuro è oggi non è uno slogan, ma una realtà che faremmo bene a cogliere anche noi che abbiamo lavorare in questa prestigiosa Aula. Signor Presidente, abbiamo parlato di responsabilità, della nostra responsabilità, di quella del Governo, delle istituzioni pubbliche. La responsabilità però non può fermarsi qui: deve coinvolgere le parti sociali e gli enti locali, e non solo. Cassa depositi e prestiti, fondazioni bancarie, importanti realtà private: costoro hanno oggi nella loro disponibilità somme rilevantissime. È questo il momento in cui anche tali soggetti sblocchino gli investimenti in infrastrutture ed energia. Non finanziamenti a pioggia o ai soliti noti; tutti dobbiamo essere guidati dalla priorità dell'interesse nazionale e questo oggi significa spendere, e spendere bene i soldi che ci sono. Responsabilità è condividere, pubblico e privato, nazionale e locale, una comune strategia di crescita e di sviluppo. Non abbiamo molto tempo: la crisi galoppa e nei prossimi mesi assumerà dimensioni davvero preoccupanti. Il Parlamento deve fare la sua parte e dare il buon esempio. Per questo mi rivolgo in modo non formale all'opposizione. a rivolgere è a non alimentare una contrapposizione di maniera sul provvedimento in esame e ad approfittare invece di questa discussione per condividere una strategia di più largo respiro. In Commissione ciò è accaduto e mi auguro davvero che prosegua anche in questa Aula.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il nostro giudizio su questa manovra cosiddetta anticrisi è di assoluta insufficienza ed inefficacia. Tale giudizio è andato vieppiù consolidandosi man mano che la crisi andava dispiegando tutti i suoi effetti negativi sull'andamento del prodotto interno lordo, sull'occupazione, sul reddito delle famiglie e sulla finanza pubblica. I fatti, ampiamente prevedibili anche alla data in discussione, ci stanno dando purtroppo ragione e la politica del Governo si manifesta sempre più inadeguata e miope di fronte a ciò che sta accadendo, ossia la più grave e prolungata crisi economica dal dopoguerra ad oggi. Spesso è accaduto in questa legislatura che il titolo, la denominazione del provvedimento fosse enfatica rispetto al contenuto effettivo delle disposizioni. In questo caso il divario tra gli obiettivi indicati e l'effettività delle misure appare ancora più di un decreto anticrisi che non inciderà in alcun modo sull'andamento della recessione in atto, ahinoi, destinata nel corso di quest'anno a subire un'ulteriore accelerazione. «La recessione è più dura del previsto. La produzione industriale scende del 13 per cento, il PIL del 2 per cento»; «stimiamo che ci saranno, nei prossimi mesi, 600.000 disoccupati in più»; «il quadro è drammaticamente cambiato»; «la politica economica è in mezzo al guado»: chi dice queste cose, onorevoli colleghi, non è l'opposizione, non sono i sindacati, non sono gli avversari di questo Governo, bensì la presidente

L'Europa, la Banca d'Italia, gli istituti di ricerca concordano nelle previsioni più pessimistiche, il che, in assenza di interventi idonei a invertire la tendenza, la tendenza, genera ulteriore sfiducia negli operatori e nelle famiglie, alimentando la spirale recessiva e il calo dei consumi soltanto attenuato dalla riduzione dell'inflazione. A fronte di tale quadro, autorevolmente certificato, come dicevo prima, sia dall'Unione europea che dalla Banca d'Italia, il Ministro dell'economia si è limitato a dire, com'è noto, che il 2 per cento in meno di PIL non è il ritorno al medioevo. Un'affermazione grave e una colpevole sottovalutazione. Non è, com'è noto, la media del calo del PIL, pur grave, che rileva, ma i fenomeni reali sottostanti. Moltissime aziende non subiscono quella riduzione media, ma una riduzione ben più consistente degli ordinativi e dell'occupazione che sta mettendo a serio rischio pezzi interi del nostro sistema produttivo e milioni di famiglie. A fronte di questa crisi, gli altri Paesi, com'è noto, stanno producendo sforzi qualitativamente e quantitativamente ben più consistenti: 73 miliardi di euro la Germania, 41 la Spagna, 26 la Francia, 24 il Regno Unito, 825 miliardi di dollari gli Stati Uniti di Barack Obama. Un intervento *shock* per quella economia, basato sull'ambiente, sulla sanità, sull'istruzione e sulle infrastrutture: quattro pilastri su cui poggia un piano energico di stimolo economico che genererà, secondo le previsioni, fino a quattro milioni di nuovi posti di lavoro. Ha dichiarato il presidente Obama: raddoppieremo la nostra capacità produttiva di energia alternativa nei prossimi tre anni (per raggiungere il livello attuale ci erano voluti 30 anni) e costruiremo una rete elettrica di quasi 5.000 chilometri, che sarà alimentata da queste nuove fonti e attraverserà tutto il Paese. Risparmieremo 2 miliardi all'anno rendendo il 75 per cento degli edifici federali più efficienti dal punto di vista energetico e le famiglie pagheranno bollette più leggere risparmiando in media 350 dollari all'anno. Questo è lo sforzo che si sta producendo nel mondo. Per quanto ci riguarda, approviamo un provvedimento come quello che stiamo discutendo, che per onestà intellettuale gli stessi relatori hanno definito superato dagli eventi e insufficiente, che reca un misero impegno finanziario di 5 miliardi di euro. Gli effetti stimati sul PIL di questo provvedimento sono di un decimo di punto e a ciò deve aggiungersi - ahinoi - il carattere fortemente restrittivo della manovra triennale di luglio (31 miliardi di euro di risorse in meno), che contribuisce ulteriormente a deprimere la nostra domanda interna, compresa quella per gli investimenti. La manovra appare inefficace a mutare l'andamento macroeconomico perché non è tale da non mutare e, per certi versi, prevede l'esatto contrario di ciò che nelle economie più colpite dalla crisi e più affini alle nostre si sta facendo. Basti pensare alla misura sull'efficienza energetica degli edifici,

sulle rate dei mutui è una misura propagandistica in una fase di forte riduzione dei tassi di interesse. La misura del *bonus* è di bassissima entità, temporanea, *una tantum* e quindi non tale da poter generare una inversione nelle aspettative delle famiglie italiane, quanto meno relativamente al soddisfacimento dei bisogni Certo, alcune delle misure contenute nel decreto appaiono di per sé condivisibili, ma ciò non muta la nostra valutazione sull'impatto complessivo dell'intervento, che - come ho detto - non non è destinato a cambiare, né ad incidere significativamente sul costo della crisi in atto e in fase di accelerazione. Abbiamo formulato le nostre proposte alternative, come abbiamo fatto

ed è così sinteticamente riassumibile: ciò che serve al nostro Paese è la riduzione della pressione fiscale sui redditi medio-bassi, quindi più reddito per le famiglie che non ce la fanno, dando in tal modo modo un impulso ai consumi, e dunque alla ripresa della nostra economia; utilizzo di un punto di PIL, con contestuale individuazione delle misure di riduzione della spesa corrente, per rientrare dallo sforamento consentito dai criteri di flessibilità previsti nel Patto di stabilità europeo a partire dal 2010. Voi insisterete ovviamente sulle vostre posizioni, asserendo la necessità primaria della stabilizzazione dei conti, che noi abbiamo sempre condiviso e che condividiamo, ma che non è antitetica alle necessità cui mi riferivo. Il rischio è che avremo ugualmente (come sta già accadendo) più deficit e più debito, senza aver contribuito a stimolare l'economia, e quindi con più recessione, più disoccupazione, meno reddito per le famiglie ed ulteriore peggioramento dei conti pubblici. Noi insisteremo e voi continuerete a non dare ascolto né a noi, né a quanti in numero

in particolare questo ramo del Parlamento, non è stato messo in condizione di discutere approfonditamente cause, rimedi ed entità delle risorse finanziarie per fronteggiare la crisi, né il complesso dei provvedimenti economici Dall'inizio della legislatura numerosi sono stati i provvedimenti economico-finanziari, ma la possibilità di intervento di questo ramo del Parlamento è stata pressoché inesistente.

intervenire per modificare questo stato di cose. Continueremo nella nostra battaglia di opposizione propositiva, convinti che prima o poi non voi, ma il Paese riconoscerà la fondatezza delle nostre analisi, delle nostre gravi preoccupazioni, delle nostre proposte.

Va allora subito sgombrato il campo da ogni equivoco: sarebbe enormemente peggio per il nostro Paese, per le fasce più deboli, se questo decreto, così com'è, non fosse Sgombrato il campo da tale equivoco, possiamo andare a valutare in quale momento questa decisione è stata assunta e a fronte di quali problematiche e prospettive.

le previsioni sull'economia internazionale, europea ed italiana erano certamente non rosee. Ricordo che, fino ad ottobre-novembre, tutti i centri internazionali, in particolare quelli europei, nonché la stessa Commissione europea e la stessa Banca centrale europea davano una crescita negativa per i

questo decreto anticrisi aveva di fronte quel tipo di scenario economico, più o meno condiviso soprattutto dalle istituzioni più importanti; d'altro canto, quel decreto aveva ed ha un altro vincolo, cioè quello di determinare, (nei limiti del possibile, al massimo possibile) un sostegno all'economia senza creare un euro in più di deficit pubblico. Allora, signor Presidente, cari colleghi, è evidente che - purtroppo - da ottobre-novembre a gennaio questo quadro di riferimento è mutato è mutato anche dal punto di vista delle convinzioni delle maggiori istituzioni europee che, peraltro, sono largamente responsabili di questo stesso quadro economico certamente non positivo.

Ciò dimostra le colpe della politica economica europea, che denuncio da tempo, ma non per il gusto di accusare gli altri, perché alla fine di questo intervento assumerò le responsabilità della politica italiana, dati quei condizionamenti.

determina la totale impotenza di fronte ad una frenata dell'economia che porta tutti i Paesi europei a sfondare il tre per cento, senza che la Commissione europea possa alzare mezzo dito. Per fortuna, il Governo italiano aveva in parte anticipato a luglio la manovra, non perché mal comune sia mezzo gaudio, ma perché la verità dei dati economici deve essere la base fondamentale di qualunque serio confronto fra maggioranza e opposizione in questo Paese, ma anche tra l'Italia e le istituzioni europee.

ciò che il mio piccolo centro studi economia reale si era permesso di indicare con analisi mai contestate da nessuno (e sarei felice se lo fossero state). Mi riferisco cioè al fatto che quella linea masochistica di politica economica europea avviene con un chiaro *trade off* di cui dobbiamo avere consapevolezza, ma che le due autorità, Banca centrale europea e Commissione europea, avrebbero dovuto comunicare con chiarezza e trasparenza ai Governi e ai cittadini europei,

Ciò detto, non ho sentito mezza parola, né in Commissione né in quest'Aula, da parte di autorevoli membri dell'opposizione - che, a mio parere, conoscono queste cose - per illustrare il quadro di riferimento nel quale il Governo italiano si trova ad operare - come altri Governi italiani - in una condizione che francamente non mi sarei aspettato.

Questo decreto, con le misure che contiene, è in grado - quantitativamente e qualitativamente - di fronteggiare la prospettiva per il 2009 di una crescita negativa del 2 a parità di condizioni di equilibrio di finanza pubblica? La risposta, collega Legnini, è banalmente «no», ma, se non passasse questo decreto, avremmo costi enormemente superiori; una maggioranza, però, deve essere consapevole dei passi che deve compiere, via via

abbiamo solo quadri di riferimento. Quindi, la risposta è «no», ma la responsabilità politica di quest'Aula è fare in modo che questo decreto venga approvato il più presto possibile, per poi aprire un confronto serio

una manovra quantitativamente forte e sufficiente a compensare in larga misura quel meno 2

quantitativamente molto più importanti che non se dovessimo approntarne per un milione e mezzo di persone. Questa è la responsabilità politica di maggioranza e opposizione al confronto e questa manovra, quantitativamente più consistente, che deve avere carattere strutturale e permanente, presenta una condizione sulla quale dobbiamo fare chiarezza: deve essere fatta senza un euro in più di deficit:

Qual è la sintesi di questa proposta? Sul piano delle quantità, si propone una manovra da 16 miliardi, pari all'1 per PIL. Mi permetto di dire che non basta neanche quello, sul piano delle quantità, perché ne occorre una seria, di due punti di PIL: 30-35 miliardi è il numero che ripeto da parecchi mesi.

minori tasse e aumenti di spesa senza dare la copertura, ma che la copertura la mettiamo nel 2010 e nel 2011, con mezzo punto nel 2010 e un punto e mezzo nel 2011. 2011. Francamente, se non vogliamo prenderci in giro, non si può proporre un giochetto del genere perché sarebbe pericolosissimo, non tanto per le procedure della Commissione europea

elemento è stato parzialmente corretto dicendo che si predispongono aumenti di tasse per cui l'effetto sul *deficit* sarebbe solo 0,4-0,5 per cento. Allora di cosa stiamo parlando?

essere forte a fronte dell'andamento del quadro di previsioni su cui concordiamo, deve essere di 30-35 miliardi e coperta, quindi senza un euro di *deficit*. Mi sono permesso di indicare le coperture,

tutti gli sperperi delle spese per acquisti delle pubbliche amministrazioni (mi rimetto alla bontà dei colleghi se vorranno leggere analiticamente l'impalcatura di questa manovra), per destinare le seguenti risorse: 15 miliardi di euro, introducendo una deduzione per carichi familiari di 5.000 euro per ogni componente del nucleo;

l'opposizione se la sente politicamente di indicare cosa tagliare, prima di dire cosa dare?

quali sono gli strumenti per sostenere famiglie, imprese ed il rilancio delle infrastrutture. Io ci ho provato avanzando una proposta provocatoria, anche nei

ci sia un qualunque rischio di sforamento dei tempi per colpa o per attività dell'opposizione, dal momento che i tempi sono contingentati e, quindi, è matematico che si voti mercoledì.

decreto-legge e fiducia, pure in una condizione che vede una maggioranza più che confortevole, e ciò finisce per diventare davvero un calpestamento totale delle prerogative parlamentari.

Proprio perché l'esercizio è questo, forse è possibile svolgere qualche ragionamento più di fondo non sulla crisi ma sulla gestione della crisi e su quello che d'ora in poi si può fare.

Non appartengo per cultura a chi pensa o pratica il «tanto peggio, tanto meglio». Penso, anzi, che di fronte a crisi di questo tipo un Paese debba essere capace di fare fronte comune. Lo dico con grande nettezza.

ciò non ci esime, cari colleghi, dal puntualizzare alcune differenze di fondo; io dirò le mie. Innanzitutto, non condivido, non ho condiviso, l'analisi della crisi mondiale anticipata nell'osannatissimo libro del ministro Tremonti «La paura e la speranza». Per mesi ci è stato detto che il pericolo arrivava dalla Cina, dall'invasione cinese, dall'errore di aver fatto entrare la Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio, attribuendolo peraltro ad una volontà della Commissione europea guidata dal presidente Prodi, all'epoca in cui il ministro Tremonti era ministro del Governo italiano (che sicuramente non ho visto sulle barricate). Certo, una distrazione geografica notevole. Non solo la crisi non è arrivata dalla Cina, oggi dobbiamo sperare e pregare che la Cina resista per mille ragioni che non voglio qui elaborare, ma che mi paiono evidenti. La crisi è arrivata da altra parte: è arrivata da Ovest

eccessivo mercatismo, dunque, ma esattamente perché mala politica ha consentito, promesso e protetto un'esposizione finanziaria dei fondi Fannie e Freddie al di là di quanto fosse concepibile.

un titolo mal posto e quanto mai altisonante. Ed anche nella gestione della crisi, di cui le istituzioni europee ci hanno avvertito in tempo - certamente non ha prodotto uno strumento non prudente, ma inadeguato e insufficiente, tant'è vero che siamo qui a discutere, giusto per occupare il tempo fino a mercoledì, augurandoci di discutere più utilmente sul prossimo

Ma a luglio cosa si è deciso? Si è deciso di spendere, sostanzialmente in termini di minore entrata, 4 miliardi di ICI.

Non voglio tornare sulla questione se non per dire che mi preoccupa un Paese in cui il Presidente del Consiglio ha la possibilità di affermare pubblicamente, che chiunque

a crisi globali si risponde con misure globali e non con misure protezioniste, nazionaliste o localiste. Inoltre, è vero che azioni vero che azioni già prese senza consultare nessuno portano sicuramente oggi il nostro Paese, che con il *deficit* che si ritrova già in difficoltà, in una posizione diversa.

Forse non è questa la preoccupazione dei cittadini italiani.

Capisco l'attacco del senatore Baldassarri, la sua critica alla politica economica della Unione europea; però dobbiamo anche riconoscere che i vincoli e le rigidità introdotte dai Trattati di Maastricht hanno garantito al nostro continente, e quindi anche all'Italia, una condizione che risulta oggi favorevole, di vantaggio, rispetto ad altri contesti, dove invece si è accumulato un eccessivo eccessivo ricorso al debito privato, a causa del quale ci troviamo di fronte ad una crisi ingovernabile.

Quindi oggi stiamo cercando di ritrovare il bandolo della matassa. Anche noi italiani abbiamo coltivato l'idea che quel liberismo

il provvedimento che riguarda la Cassa depositi e prestiti è un articoletto inserito senza grandi spiegazioni. In realtà si tratta di un'ulteriore liberalizzazione; ulteriore perché, già con la riforma del 2003 (ma ancor prima con i provvedimenti approvati nel 1992, che cancellavano il contributo a carico dello Stato per sostenere gli investimenti degli enti locali),

oggi - il caso di Milano è solo uno ed è forse la punta dell'*iceberg* - che gli accordi sui derivati fatti dagli enti locali nascondono l'incrocio tra

Oggi ci accorgiamo che nessuno è in grado di stabilire la massa di queste operazioni finanziarie, forse con qualche problema di corruzione

davvero uno dei possibili fulcri di una grande manovra finanziaria, il Parlamento deve affrontarlo con organicità e con serietà e non in questa maniera.

Debito pubblico: il differenziale del rendimento sulle scadenze decennali di riferimento ha toccato il massimo dall'introduzione dell'euro, a 157 punti base Libertà economica: Italia a picco nella classifica del «Wall Street Journal», siamo al 76° posto, peggio del Kirghizistan; in un anno abbiamo perso dodici posizioni. Disoccupazione: le organizzazioni degli imprenditori stimano la perdita di 600.000 posti di lavoro; le organizzazioni sindacali arrivano a stimarne più di 1.000.000; imprese storiche chiuderanno i battenti. Consumatori: scende a picco la fiducia del consumatori che vedono nero nel loro futuro. In merito alle banche, mentre il Governo afferma che le banche italiane stanno meglio delle altre,

E mentre il pianeta va incontro ad una delle più gravi crisi economiche, ben superiore a quella del 1929 per gli effetti della globalizzazione (una crisi provocata dalla creazione del denaro dal nulla, dall'avidità dei banchieri che il Governo salva, dalla collusione delle agenzie di *rating* e dalla complicità delle banche centrali); mentre inascoltate Cassandre denunciavano gli effetti di una gravissima crisi finanziaria, che sta mangiando l'economia reale con la perdita dei posti di lavoro, soprattutto nell'Italia dei cartelli, dei monopoli e delle corporazioni (coadiuvate dal Governo che ha rimandato alle calende greche la *class action*); mentre i Paesi importanti, a cominciare da Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Spagna e Cina, varano misure anticicliche ed assumono impegni seri per nuovi investimenti pubblici, pari a circa 7 punti del PIL, la strategia dell'Italia per fronteggiare la crisi non arriva neppure allo 0,3 per Allora, o il Governo, nella famigerata manovra di giugno approvata nel Consiglio dei ministri in meno di nove minuti, non aveva intuito la gravità della crisi, oppure, se aveva letto nella palla di vetro del futuro, non doveva approvare un vero e proprio sperpero di pubblico denaro, quantificato in ben 7 miliardi di euro (tra i 4 miliardi accollati alla fiscalità generale per Alitalia e l'abolizione dell'ICI, non nei confronti delle prime case, ma di chi non ne aveva bisogno). Ho già avuto occasione di soffermarmi in Commissione sul fatto che il Governo non ha ancora oggi la diretta percezione di una crisi che viene da lontano; ha paragonato questa manovrina anticrisi alle stregua del gioco delle tre carte di collaudati prestigiatori, una manovra piena di illusioni e priva di effetti reali sulle famiglie e sulle imprese. Ci sono somme che vengono e vanno: sono spostate con la stessa rapidità del mago Silvan da una posta all'altra del bilancio dello Stato. Voglio ricordare che il 16 novembre scorso a Washington, il ministro Tremonti, forse contagiato da Barack Obama, annunciò un piano roboante da 80 miliardi di euro. Dopo soli tre giorni quei miliardi diventarono 12,7, per scendere poi a 7, a 6,5 ed infine, il 29 novembre, a 3,7 miliardi. Oggi ci ritroviamo ad avere un intervento a saldo zero; più precisamente, il decreto anticrisi ha un saldo netto in positivo, tra variazioni nette nelle entrate e nelle uscite, di 390 milioni Non solo non c'è una riduzione della pressione fiscale, ma vi è un incremento netto delle entrate, in gran parte tributarie, di 3 miliardi e mezzo che serve più che a compensare l'aumento netto delle spese. L'aggressione al potere d'acquisto di lavoratori e pensionati viene da lontano: dalla gestione del *changeover*, che ha scientemente permesso alla speculazione sui prezzi al consumo di galoppare a briglia sciolta, mentre l'erogazione di salari e pensioni è avvenuta con rigorosa corrispondenza rispetto alle vecchie lire. Tale aggressione si è avvalsa anche della politica fiscale, che, mentre favoriva ricchi ed evasori (ricordiamo ancora lo scudo fiscale del ministro Tremonti), colpiva i redditi medio-bassi con la mancata restituzione del *fiscal drag*. si è avvalsa della consapevole manipolazione dei criteri di determinazione delle retribuzioni, attuata attraverso la fissazione di tassi di inflazione programmata sistematicamente ed ampiamente inferiori all'inflazione reale.

tale pacatezza non corrisponde alla coscienza di questa crisi perché questo decreto anticrisi ha un saldo netto in positivo di 390 milioni e, quindi, le misure di spesa appaiono sottofinanziate. Per esempio, la *social card* - la "umilia *card*", com'è stata ribattezzata - costerà più di quanto è stato appostato nel bilancio. Il *deficit* lasciato dal precedente Governo era al di sotto del 2 per cento. A metà novembre, cioè prima della manovra approvata venerdì scorso ma dopo la finanziaria 2009, il *deficit* viaggiava attorno al 3 Scontava, infatti, come ho detto: i 3 miliardi dovuti all'abolizione dell'ICI; i 3 miliardi versati ai "capitani coraggiosi" per l'Alitalia; l'aumento del fabbisogno derivante dai minori incassi tributari. L'insieme di queste misure ha peggiorato i nostri conti pubblici. Per questo abbiamo parlato di vero e proprio sperpero di risorse: quei 7 miliardi avrebbero fatto molto comodo oggi. Mi dispiace che il presidente Baldassarri non abbia ascoltato

le mani. Anche sul punto abbiamo assunto una posizione molto critica. Noi avevamo proposto di tagliare gli sprechi e devolverli al sostegno duraturo dei salari, cioè ad una vera e propria redistribuzione del reddito; tassare i redditi miliardari, le innumerevoli rendite esistenti, i redditi sommersi; di puntare sulla crescita e sulle nuove risorse tributarie che essa determinerebbe.

Questo dovrebbe valere per tutti; noi però ci atteniamo. L'intervento sui mutui (sulla commissione sul massimo scoperto stendo un velo pietoso) è il riconoscimento del fallimento,

e dispone che le banche offrano contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato al tasso di rifinanziamento principale della BCE in alternativa all'Euribor, (che oggi ha raggiunto il minimo storico del 2,15 Il ritardo del Governo implica un costo di diverse centinaia di euro per le famiglie con mutui a tasso variabile. In ogni caso, va sottolineato che gli oneri per i minori interessi pagati dalle famiglie saranno a carico del bilancio dello Stato. Ancora una volta, nessun sostegno per i mutuatari a tassi fissi, nessun impulso alla competizione tra aziende di credito e nessun sostegno al meccanismo della portabilità dei mutui.

non si va a vedere che i soldi li dovrebbero dare alle piccole e medie imprese, e si salvano i bancarottieri. È una cosa per noi scandalosa. Signora Presidente, la crisi sta dimostrando giorno dopo giorno di affondare le sue radici nell'economia reale. Ciò porta gli analisti e i centri di ricerca, soprattutto quelli che godono di maggiore fiducia nel panorama internazionale, a non prevederne tempi e confini. È certo oramai che la recessione in corso presenti aspetti molto forti e consistenti, tali da evidenziare il sicuro rischio di preoccupanti effetti negativi sul reddito e sull'occupazione. Tutto ciò richiederebbe una discussione ampia e partecipata, in grado di mettere al centro, a mio avviso, politiche e misure volte a determinare la ripresa della crescita e il superamento di vecchie e nuove sperequazioni che gravano pesantemente sul nostro sistema Paese. situazioni che, se non affrontate con lungimiranza proprio in questa fase così difficile, possono determinare ulteriori gravi diseguaglianze e ritardi nell'ammodernamento del Paese. Da questo punto di vista, non si tratta di scegliere tra ottimismo e pessimismo, ma piuttosto di considerare in modo serio e preciso gli effetti che già ora la recessione manifesta in termini di tenuta economica e sociale del Paese, prevedendo al contempo la messa in campo di risposte in grado di offrire a tutti i soggetti economici e sociali una possibile via d'uscita, in un quadro di maggiore efficienza del sistema e di migliori condizioni di coesione sociale. Su questo versante si muove, a mio avviso, la proposta avanzata dal Gruppo PD, prima nella discussione sulla finanziaria e oggi sul decreto anticrisi. Attenzione particolare viene data e, in via prioritaria, agli effetti della recessione sul fronte dell'occupazione, del lavoro. Già oggi i dati ci dicono che circa 500.000 lavoratori sono posti in cassa integrazione, e che per un milione di precari esiste il rischio del mancato rinnovo. È una grande questione sociale, che deve spronare la politica, direi tutta la collettività nazionale, a riaffermare dentro la crisi nuove frontiere di solidarietà. Su questo crinale si colloca la consapevolezza che garantire il reddito dei nuovi disoccupati, soprattutto per chi non è coperto da alcuna protezione, può certo servire a sostenere i consumi, ma soprattutto mira a dare un segno di solidarietà a chi viene colpito dalla crisi. In tal modo, inoltre, si può salvaguardare un capitale umano e sociale di straordinarie dimensioni, un capitale che, rimanendo inalterato, può offrire il giusto contributo allo sviluppo del Paese. Nella crisi del 1992-1994 andarono perduti circa 1.400.000 posti di lavori. Ora deve sorgere in noi la consapevolezza che, diversamente da allora, la quota di nuovi disoccupati garantiti da strumenti di sostegno, in particolare i prepensionamenti, sarà molto più bassa, perché l'attuale mercato del lavoro è composto da ampie fasce di lavoratori non protetti, soprattutto giovani e perciò non prepensionabili. È necessario, quindi, un nuovo quadro di ammortizzatori sociali a carattere universalistico proprio a partire dall'introduzione di misure di sostegno al reddito di quei disoccupati sprovvisti di copertura assicurativa, associando tutto ciò all'attività di formazione e programmi di reinserimento lavorativo. Va data quindi grande attenzione alla condizione dei lavoratori, a partire dai giovani, dai precari. In questo quadro si inserisce, in modo magari non diretto, ma in ogni caso meritevole di attenzione, un punto del provvedimento in esame che riguarda le condizioni di precarietà di molti nostri connazionali giovani in servizio nelle Forze armate. Infatti, anche a seguito delle giuste proteste dei lavoratori del comparto difesa e sicurezza per i tagli indiscriminati apportati a quel settore, la maggioranza ha previsto in via sperimentale che al personale del comparto titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore nell'anno 2008 a 35.000 euro venga riconosciuta una defiscalizzazione sul trattamento economico. È una misura molto limitata: si tratta di circa 150 euro *pro capite*. Tale misura, però, non sarà applicabile a circa 32.000 militari, oggi volontari in ferma annuale e in ferma breve, perché percettori non di uno stipendio ma di una paga giornaliera. Questi "precari" delle Forze armate sono i più giovani in servizio e sono il serbatoio che alimenta, in termini di personale, le missioni internazionali all'estero e quei compiti di ordine pubblico, affidati alle Forze armate, in ragione anche delle ultime decisioni assunte dal Governo. Ci attenderemmo, quindi, una maggiore attenzione da parte della maggioranza per quei lavoratori precari alle dirette dipendenze dello Stato, impiegati, oltre tutto, in particolari e delicatissimi scenari operativi. Quest'ultima considerazione, signora Presidente, mi permette infine, rimanendo nel comparto difesa e sicurezza, di affermare che i necessari interventi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica in questo settore trovano questa parte politica assolutamente disponibile al confronto di merito. È certo, però, che di questo si dovrà trattare. Non mi pare, invece, che così si muovano il Governo e la maggioranza: prima operano tagli indiscriminati nel settore della difesa senza un quadro strategico di riferimento e poi, invece, intendono realizzare consistenti spese per sostenere interventi quali quelli annunciati in queste ore, che risultano, oltre che discutibili nel merito, anche particolarmente costosi. In questo frangente, sarebbe meglio agire con decisione sul fronte dell'assegnazione di adeguate risorse al settore dell'ordine pubblico, operando al contempo, come detto, una meticolosa e seria razionalizzazione della spesa di tutto il comparto difesa e sicurezza. È solo questione di volontà politica e noi siamo pronti a perseguirla, anche perché sappiamo che da questo quadro e da questo processo di razionalizzazione possono scaturire quei miglioramenti allo stato generale della spesa pubblica capaci di coprire, nei prossimi anni, la manovra espansiva di cui oggi il Paese necessita.

la crisi finanziaria, iniziata nell'agosto 2007 negli USA, è dilagata velocemente, diventando inevitabilmente crisi sistemica e planetaria. Essa porta con sé la fine di un certo modello di economia che ha stravolto i ruoli degli attori economici: banche e società finanziarie in primo luogo, ma anche imprese, Governi e risparmiatori. I dati ISTAT relativi al settore industriale italiano dicono che, rispetto ad un anno fa, il fatturato è diminuito del 13,9 per cento, mentre il calo degli ordinativi ha toccato il 26,2 per un crollo della domanda interna e degli investimenti che minaccia, nel medio periodo, i livelli occupazionali. La crisi non ha esaurito il proprio potenziale distruttivo di ricchezza, e gli analisti, pur con previsioni discordi, ritengono che durerà ancora. Diamo dunque atto al Governo italiano di essere stato, già dal mese di luglio, forse il primo - anzi, in Europa sicuramente il primo - a mettere in campo misure importanti a sostegno sia delle famiglie che delle imprese. Ciò, nel rispetto di un obiettivo vitale: garantire che entro il 2011 il debito pubblico scenda sotto il 100 per Un traguardo necessario per consolidare la fiducia degli investitori nei confronti dell'Italia e per sanare la grave situazione dei nostri conti pubblici, dei quali non dobbiamo mai dimenticare l'importanza. L'azione italiana è stata poi seguita, più tardi, dal piano dell'Unione europea per l'uscita dalla crisi: i 27 Paesi dell'Unione si sono accordati su una manovra congiunturale a sostegno dell'economia reale che prevede un incentivo finanziario coordinato pari a circa 200 miliardi di euro (1,5 per cento del PIL), a livello nazionale,

Mi riferisco, per esempio (e ritengo questo aspetto molto importante, provenendo dalla Commissione lavoro), agli 8 miliardi di euro stanziati per gli ammortizzatori sociali e l'ampliamento della platea degli aventi diritto che oggi ricomprende i lavoratori che non hanno un lavoro stabile e le aziende più piccole: sono dunque ammortizzatori

Il decreto che stiamo esaminando è dunque parte di un'azione più vasta e complessa, che rappresenta il massimo di quanto ci è consentito con le risorse a disposizione e con il debito - tema sul quale ritorno - che ha il nostro Paese.

poggia su due pilastri: il sostegno alle famiglie, con il conseguente rilancio della domanda interna, e il sostegno alle attività produttive, per offrire possibilità di crescita economica. II sostegno alle famiglie si basa soprattutto sul *bonus*, che da solo vale 2,4 miliardi di euro, e sulla detassazione dei premi di produttività per i lavoratori, per un impegno di ulteriori 400 milioni di euro. Per le imprese è prevista la deducibilità del 10 per cento dell'IRAP su IRPEF ed IRES, per sgravi complessivi di circa 1,2 miliardi di euro. Non dimentichiamo poi l'IVA differita

concentrato su queste due azioni, in modo da rendere più incisivi gli effetti sul sistema economico. Non manca tuttavia una serie di provvedimenti che non sono arrivati alle cronache dei giornali, ma che sono importanti.

che vengono congelate per un anno o per le quali si prevede un ampliamento delle fasce sociali. Discorso a parte merita il fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato (che mi sta particolarmente a cuore, esposto

Il potenziamento del trasporto su rotaia, poi, con una mole di investimenti notevole, può essere un volano importante per lo sviluppo. Completa tale strategia l'autorizzazione ad una spesa di 480 milioni di euro all'anno, per tre anni, per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato, Regioni e Trenitalia spa (e ciò coinvolge i nostri pendolari). L'erogazione delle somme è condizionata anche al fatto che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, come accennavo anche prima. Questa è indubbiamente una buona notizia,

sulla base dei contratti stipulati dalle Regioni con Trenitalia spa, anche dei diritti dei cittadini che vivono nelle zone meno servite dal gruppo Ferrovie dello Stato. Sarebbe davvero inconcepibile che, volendo dare slancio alla mobilità su rotaia, si permettesse una gestione residuale di questi utenti, che rischiano di essere tagliati fuori dal trasporto veloce, in generale, e dagli Eurostar, in particolare. Ho visto che si punta molto e si scommette sull'Alta velocità, ma l'Italia è lunga e ha bisogno di linee di trasporto.

l'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale, riducendo le sanzioni applicabili. Si esce dunque dall'ottica dello Stato che sa solo punire e secondo le previsioni questo dovrebbe far salire le entrate di quasi 145 milioni di euro (e speriamo che questo accada veramente). Degna di nota è la lotta all'evasione, attuata con il maggiore controllo fiscale per le imprese di più rilevante dimensione, quelle cioè che conseguono un volume di affari e ricavi non inferiore a 300 milioni di euro. Tale importo verrà gradatamente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, per queste aziende i controlli sostanziali saranno continui.

significa che non si doveva intervenire, come si è giustamente fatto e si sta facendo ancora con determinazione, soprattutto a sostegno delle realtà più deboli ed esposte.

significa intraprendere, creare e dare lavoro: è forse grazie a questa sua capacità, che non è solo politica ma si tocca con mano, che possiamo affrontare i tanti problemi che assalgono adesso il Paese.

oggi apriamo e chiudiamo in poche ore la discussione sul decreto-legge n. 185, che ridisegna in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale; oggi insomma stiamo discutendo la strategia del Governo della Repubblica per fronteggiare la crisi del secolo.

una situazione in cui in poco più di undici mesi sono stati spazzati 25.000 miliardi di dollari dai listini delle borse mondiali

in queste poche ore - e tra pochi - in risposta alla crisi del secolo. È un dato che mi lascia veramente perplessa, mi lascia veramente perplessa, perché considero che in quest'Aula abbiamo dedicato più tempo, in proporzione, a discutere delle corse dei cavalli, dei giochi e dei finanziamenti a questo settore che non

a tutto questo non si è arrivati e vi è stata una dispersione di potenzialità del Senato della Repubblica che credo non torni a nostro vantaggio. rileggerà la crisi del secolo e, andando a cercare quali sono stati gli atti con cui il Parlamento della Repubblica vi ha risposto, troverà questo come decreto anticrisi - testualmente - «per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale». dovendo cercare gli elementi messi in campo per rispondere alla crisi, troverà articoli sulle addizionali sulla produzione e vendita di materiale pornografico, sull'IVA dei documenti di viaggio nei trasporti pubblici urbani e anche qualcosa sui parcheggi veicolari. In questo, che difficilmente riesco ad immaginare come strumento strategico per combattere la crisi, dovrà trovare la nostra politica per combattere la crisi del secolo, che pure c'è, è cattiva, brutale e, sicuramente, lunga. È cattiva perché la sua genesi è del tutto particolare, rispetto a quelle che l'hanno preceduta, ed è difficile da codificare. È brutale, perché negli Stati Uniti si sono già persi 1,7 milioni di posti di lavoro e da

degli Stati. Sarà quindi importante che ogni Stato sappia come giungere alla fine della crisi (che certamente finirà) in condizioni tali da agganciare la ripresa. credo che all'interno di questo documento non vi siano gli elementi che consentano di fare questo, ossia essere pronti, alla chiusura della crisi, ad agganciare la ripresa, che senz'altro ci sarà.

l'elemento strategico per consentire al nostro Paese di uscire in termini positivi da questa crisi è quello di rafforzare le azioni a sostegno delle piccole e medie imprese. Sei milioni

i tanti rivoli, in cui comunque molta spesa è stata diluita, concentrarli in una sola operazione e, a questo riguardo, compierne una decisa, rispetto a questo solo, singolo punto nei confronti delle piccole e medie imprese, chiudendo questa pagina indecente dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Si sarebbe potuto fare, raccogliendo evidentemente risorse diversamente utilizzate in piccoli rivoli, che non producono la massa critica necessaria per risolvere problemi strutturali a questo che è un settore strategico. *(Richiami del Presidente)*. Concludo, come lei mi invita a fare, signora Presidente, dicendo solo un'ultima cosa:

la paura della crisi. La paura è una forte componente della crisi, ma non si può pensare che basti un provvedimento come questo (che è di gestione della paura della crisi), tardando

che porta un titolo molto importante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale». Mi chiedo in quali parti di questo provvedimento vi sia una qualunque lontanissima coerenza con il titolo e con le aspirazioni a cui esso vuole tendere. Come tutti abbiamo avuto modo di ricordare, stiamo attraversando una crisi non soltanto molto grave, la più grave che certamente dal dopoguerra il mondo occidentale - e adesso tutto il mondo - sta vivendo, stiamo anche attraversando una crisi il cui portato, la cui dimensione, le cui ragioni non sono in fondo ancora del tutto bene esplicitate e ancora del tutto chiarite. È una crisi che nasce per un dissesto in una parte specifica del mondo delle transazioni finanziarie, che si è già ampiamente trasferita - non che si trasferirà - sull'economia reale, che fa sentire il proprio peso in termini di recessione economica, quella prevista, quella che purtroppo osservatori più pessimisti ma di rango internazionale, come il Fondo monetario internazionale oppure l'OCSE, prevedono ancora di dimensione maggiore per l'Europa e soprattutto per un Paese come l'Italia. Siamo in una situazione in cui molti paventano che la prossima estate avremo contemporaneamente alla recessione una situazione di deflazione, che è una delle patologie più gravi da curare. Ben si ricordano di questo gli economisti che si trovarono ad affrontarla nel periodo *post* 1929, in una situazione non globalizzata ma ancora molto circoscritta. Le condizioni che si determinarono dopo la crisi del 1929 penso di non doverle richiamare, sono note a tutti. Quella crisi ha avuto degli esiti nefasti perché le politiche che sono state messe in campo per affrontarla o erano inadeguate o erano insufficienti o erano sbagliate. Questa volta non ce lo possiamo permettere. Abbiamo bisogno di esaminare, anche come Parlamento della Repubblica, una proposta finalmente realistica, organica, un'idea non catatonica della crisi, come sta dimostrando il Governo, ma un'idea complessiva su come affrontare, come Paese a forte indebitamente pubblico ma con prerogative molto positive come quelle di avere un tessuto diffuso di impresa

per il Governo, perché è una proposta esagerata e non ha le coperture; non va bene per il presidente Baldassarri, perché invece è una proposta timida e dovrebbe essere raddoppiata. Per l'amor di Dio, si può dire qualunque cosa, ma qualche proposta il Governo ha il dovere di farla; qualche proposta su come si fa una politica anticiclica e antirecessiva, agendo sul mercato interno, è necessario metterla in campo. In secondo luogo, siamo di fronte ad una recessione, cioè ad un calo della domanda, che è internazionale ma è anche interna, e le imprese, quelle piccole e piccolissime imprese che peraltro vengono solo tangenzialmente toccate da qualche marginale provvedimento (ricordo, per esempio, che il calo fiscale che viene previsto dal provvedimento in

conseguente al *credit crunch*, ma a dover fare da banca tre volte: fanno da banca verso la propria banca, perché viene richiesto a tutte le piccole imprese italiane il ritorno dagli extrafidi; fanno da banca verso i propri committenti, perché stanno gestendo il magazzino e avranno pagamenti a 180 giorni o a 240 giorni dai propri committenti ed è prendere o lasciare; stanno facendo da banca allo Stato, il quale si guarda bene dal pagare i propri debiti e dal fare una delle poche cose che si potrebbero fare rapidamente senza alterare i soldi pubblici, cioè semplicemente pagare i propri fornitori nei tempi in cui dovrebbero essere pagati. Sono manovre antirecessive. Richiederebbero altro, ma credo che in una fase come questa la cosa migliore e più necessaria da fare è sapere che alla recessione, che noi vediamo esplicarsi con numeri freddi,

Pertanto, la prima cosa che va messa in campo con molta energia e determinazione, prima ancora del sostegno alla domanda, è il sostegno a coloro che perdono il lavoro, attuando dispositivi, ammortizzatori sociali, meccanismi, anche con rapidi finanziamenti e rapide riforme, che consentano a coloro che stanno per perdere il lavoro o che sono nella condizione di perderlo, siano essi lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, di avere, in una fase

verso i mercati che debbono essere aperti, in modo che dalla concorrenza anche noi possiamo trarre qualche vantaggio che, invece, nel corso di questi anni non si è riusciti ad ottenere. Per fare questo occorrerebbe una soluzione di emergenza, un confronto politico di emergenza. Non occorrono né le filosofie del ministro Tremonti e neanche l'ottimismo di maniera del Presidente del Consiglio. Occorre non il dialogo, termine che piace poco anche a me, ma il confronto, il confronto delle idee fra le parti sociali, il Parlamento, il Governo, i *media* e l'opinione pubblica. Solo in questo modo una grande democrazia moderna può salvaguardare la propria essenza, che è essenza di informazione, di mercato che funziona, di protezione sociale e, contemporaneamente, di concorrenza. Sarebbe utile che il Governo se ne occupasse adesso, dopo il titolo ridondante riportato in questo quasi inutile fascicolo, mettendo in campo una manovra effettivamente per l'emergenza, per la crisi e cercando di trovare un vero consenso nazionale.

onorevoli colleghi, giunge all'esame dell'Aula del Senato, dopo il voto della Camera e l'approfondimento in sede di Commissioni, il decreto-legge che il Governo ha varato a fine novembre scorso con un pacchetto di misure definite anticrisi di immediata applicazione, con iniziative ed attività di sostegno alle famiglie, all'occupazione ed alle imprese. Tale provvedimento si colloca nel quadro delle misure già varate dall'Esecutivo, a cominciare dal decreto-legge n. 93 dello scorso dello scorso anno in cui si anticipavano numerose misure tradizionalmente affidate alla legge finanziaria per giungere poi nell'autunno ai provvedimenti legati alla sessione di bilancio. Si tratta, dunque, di un complesso organico di politiche che hanno dato via via risposte concrete ai bisogni ed alle necessità espresse dai cittadini e dalle imprese per far fronte ad un evento eccezionale, di eccezionale gravità e profondità, come si è rivelata essere la crisi inizialmente solo finanziaria - si riteneva - che ha colpito l'economia a livello internazionale. In tale quadro, il decreto-legge n. 185, esaminato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è uno strumento utile sia per dare una risposta immediata, ad esempio con l'istituzione del *bonus* per le famiglie a basso reddito di pronta realizzazione, sia per raccogliere le indicazioni, i suggerimenti, le proposte avanzate da più parti e inserite nel corso dell'*iter* parlamentare a Montecitorio come elemento di rafforzamento delle misure, anche adeguandole alla continua evoluzione della congiuntura socio-economica. L'estensione e l'eccezionalità della crisi in atto richiede, infatti, di poter disporre di strumenti flessibili in grado di essere via via modulati sulla base dei cambiamenti originati dall'evolversi della crisi e dalle risposte che vengono dagli altri Paesi europei e non, cercando di inquadrare le iniziative intraprese a livello nazionale con quelle che giungono dall'esterno. Il decreto-legge in esame presenta sostanzialmente due tipologie di misure. La prima è volta a dare risposte immediate per fronteggiare le difficoltà che colpiscono soprattutto le fasce sociali più deboli in modo da assicurare che le famiglie a rischio non vengano sospinte oltre la fascia della povertà con il rischio di provocare ulteriori problemi di natura sociale che potrebbero ripercuotersi sulla coesione dell'intera comunità nazionale. La seconda è costituita da iniziative che guardano più direttamente al mondo del lavoro e dell'impresa con l'obiettivo di trarre dalle sfide della crisi quelle opportunità, altrimenti difficili da conseguire, che consentano di preparare l'economia italiana a una più pronta ripresa quando la fase più acuta sarà finalmente superata e il clima internazionale consentirà finalmente di riprendere il cammino di sviluppo. Non voglio soffermarmi sul complesso di misure contenute nel decreto ed arricchite nel corso dell'esame alla Camera se non per richiamare brevemente alcuni aspetti che giudico particolarmente significativi. In primo luogo, è stata resa strutturale la decisione, in attesa del via libera delle autorità europee, dell'applicazione per il triennio 2009-2011 del regime IVA a esigibilità differita, ovvero con il criterio di pagamento per cassa anziché per competenza. Si tratta di una misura di particolare significato contenuta nel programma elettorale della coalizione che sostiene il Governo Berlusconi ed importante soprattutto per il settore delle piccole e medie imprese della subfornitura. È dunque un'iniziativa che oltre ad avere benefici immediati, nell'attuale situazione di restrizione del credito e crisi di liquidità che colpisce il mondo produttivo, trasferirà i suoi benefici effetti anche nel futuro, auspicando che quanto prima l'Unione europea conceda l'autorizzazione ad applicare questo nuovo criterio. Un secondo intervento che desidero ricordare, anche come esemplificazione di un impegno del Governo in questa direzione, è la modifica ai criteri di utilizzo del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile con l'innalzamento dell'età limite per accedere ai finanziamenti agevolati a 35 anni, l'istituzione di un fondo unico (anziché i tre attuali) e l'eliminazione di specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie d'interventi, con la conseguente maggior snellezza e semplificazione. Da ultimo, nel non esaustivo richiamo alle misure più rilevanti, desidero citare la soppressione della Commissione bancaria di massimo scoperto, se il saldo a debito per il cliente si protrae non oltre i 30 giorni, o in caso di utilizzi in assenza di fido. Si pone così termine ad una pratica anacronistica e forse anche vessatoria degli istituti di credito verso la clientela, peraltro oggetto di molti interventi già nei provvedimenti di luglio. voluto citare questi esempi anche perché comportano poca o nessuna spesa per le casse pubbliche determinando, al contrario, un beneficio immediato e rilevante per i cittadini, le imprese, gli operatori economici, ciò in linea con l'impostazione del Governo di non mettere a repentaglio i conti dello Stato, pur considerando la necessità di intervenire a sostegno dell'economia in questo delicato frangente. Infatti, la solidità e la stabilizzazione dei saldi di bilancio, la rigorosa attenzione alla gestione della finanza pubblica indubbiamente rappresentano un prerequisito su cui si basa la solidità dell'intero sistema nazionale. Pregiudicando il primo per venire in soccorso all'economia con manovre massicce che comportano un alto esborso di risorse pubbliche, si minerebbe irrimediabilmente tale presupposto. Reputo dunque più che giustificato e importante che il Governo abbia mantenuto questa linea prudenziale, resistendo alle pulsioni demagogiche e alla richiesta di talune forze politiche d'opposizione, che chiedevano forme di intervento molto più onerose. La situazione del debito pubblico italiano, appare quasi superfluo ricordarlo, non è tale da consentire al nostro Paese di affrontare iniziative che comportino un ulteriore massiccio indebitamento, pena la perdita di fiducia e di credibilità nei confronti degli investitori e dei mercati finanziari internazionali. Ciò restringe indubbiamente i margini operativi entro cui il Governo è chiamato a muoversi e rende necessario calibrare con accortezza ogni iniziativa di politica economica, valutando non solo il rapporto costi-benefici, ma anche l'impatto sul debito pubblico, con le ricadute sul *rating* del Paese. Pur nei limiti dei paletti che il Ministro dell'economia ha voluto giustamente mantenere rigidi, le misure contenute nel decreto-legge n. come negli altri atti emanati dal Governo e sanzionati dal Parlamento, hanno la caratteristica di essere iniziative puntuali, specifiche e, dalle prime valutazioni, efficaci. Un aumento non calibrato della spesa pubblica, oltre alle controindicazioni sul debito, non avrebbe del resto avuto alcuna garanzia di produrre di per sé un aumento della spesa delle famiglie, essendo legato anche al grado di fiducia esposto dai cittadini. Attualmente, tale livello di fiducia, non solo in Italia, è a livelli minimi, per la preoccupazione nei confronti degli effetti della crisi. Un aumento eccessivo delle risorse destinate a finalità sociali avrebbe potuto produrre effetti di tesaurizzazione, senza alcun beneficio per i consumi. Senza contare che, per il grado di apertura della nostra economia, una quota rilevante degli acquisti avrebbe inciso sui beni di importazione, senza benefici per le aziende nazionali. Questa è una considerazione che dovrà essere fatta anche in merito al tavolo che si aprirà nei prossimi giorni sulla crisi del settore automobilistico,

Si deve inoltre rilevare come la situazione italiana sia significativamente meno debole di quella di altre economie, a cominciare dal minore coinvolgimento dei nostri istituti bancari nei fenomeni speculativi, nella gestione dei derivati e di tutti gli strumenti finanziari oggi sotto accusa per la loro rischiosità e spregiudicatezza. Quello che era apparso - e in effetti è, in periodi normali - un segnale di debolezza del sistema bancario italiano, ovvero l'esclusione dal circuito della grande finanza internazionale, con poche eccezioni, è diventato, in un periodo di difficoltà, una forma di riparo contro le più esasperate speculazioni finanziarie. In Italia, a differenza che in altri Paesi, come ad esempio in Spagna, a fronte del pesante *stock* di debito pubblico, esiste un buon livello di patrimonializzazione delle famiglie, alimentata dalla elevata propensione al risparmio e consolidata dalla circostanza che vede le famiglie italiane in larga parte proprietarie della propria abitazione. Ciò fornisce elementi di equilibrio anche al comparto immobiliare, che in altri Paesi ha subito crolli pesanti, come non è avvenuto in Italia. In conclusione, signora Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che le misure contenute nel decreto-legge n. 185, con le integrazioni che la Camera di deputati ha saputo e potuto introdurre, siano adeguate a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie italiane e a dare supporto alle fasce deboli a rischio povertà, a stimolare l'attività produttiva, a contenere i rischi di disoccupazione, in una parola a sostenere lo sforzo dell'intero Paese in questo pur difficile frangente, costruendo le condizioni per una prossima ripresa, in attesa che l'economa internazionale possa riconquistare il segno positivo. *(Applausi

Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è una manovra sbagliata, in ritardo, incerta. Basterebbe questo per definire la manovra che stiamo discutendo. È sbagliata perché, a fronte della crisi finanziaria ed economica che il nostro Paese ed il mondo intero stanno attraversando, di ben altro si avrebbe bisogno. Mentre il Presidente degli Stati Uniti d'America, appena insediato, mette in campo una manovra anticiclica di oltre 800 miliardi di dollari, e su questa linea si muovono i principali *leader* europei, da Sarkozy alla Merkel, da noi l'Esecutivo sembra l'ultimo paladino del contenimento della spesa ed evita di dare risposte convincenti a livello della crisi. Anzi, le iniziative assunte vanno nella direzione opposta: come l'abolizione dell'ICI per i redditi più alti, le regalie per la vicenda Alitalia, i tagli indiscriminati a carattere lineare e l'abbandono della lotta all'evasione e all'elusione fiscale, che registrano anzi, stando ai dati ultimamente diffusi, un considerevole incremento. D'altronde, i dati sulla crisi, purtroppo, ogni giorno che passa, diventano sempre più allarmanti. L'ultimo bollettino economico della Banca d'Italia, confermando di fatto le analisi diffuse da Confindustria, dal Consiglio europeo e dalle organizzazioni sindacali, evidenzia che nel terzo trimestre 2008 il PIL è diminuito del 2 per cento, in conseguenza della stagnazione dei consumi, del calo delle esportazioni e delle importazioni, dei mancati investimenti delle aziende. I dati più recenti sulla disoccupazione ci riportano indietro di più di vent'anni. Recentemente la Confindustria ha elaborato degli studi che configurano gli anni 2008 e 2009 come due anni di recessione, ipotizzando una perdita di 600.000 posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione che salirà all'8,4 per cento. Siamo in presenza di un incremento vertiginoso delle richieste per cassa integrazione sia ordinaria quanto straordinaria e con l'espulsione dal mondo del lavoro di centinaia di migliaia di precari, le prime vittime di questa crisi che affrontano questa tragedia in totale assenza di qualunque tipo di rete sociale. Sembra francamente paradossale ricordare che solamente fino a pochi mesi fa l'Esecutivo era impegnato a reperire risorse per la detassazione degli straordinari. Sarebbe bene che ammetteste di aver sbagliato ogni tipo di previsione. Fate marcia indietro, cambiate strada, mettete in campo misure reali per dare risposte convincenti alla famiglie, ai lavoratori, ai pensionati e a partire dai lavoratori precari. L'*una tantum* del 10 per cento sul reddito dell'anno precedente per i precari è una misura tanto inadeguata se commisurata al reddito di questi lavoratori, in media 8.000 euro annui. Il *bonus* quindi destinerà in media a questi lavoratori 800 euro per sopravvivere alla crisi. In particolare, per questi ultimi, l'intervento obbligatorio degli enti bilaterali, così come previsto dal testo, rischia di restringere la platea dei beneficiari. Ancora misure del tutto inadeguate, come la tanto reclamizzata *social card* che doveva interessare 1.300.000 anziani, e che tra imbarazzi e umiliazioni ad oggi è stata utilizzata da soli 420.000 cittadini italiani a fronte delle 580.000 richieste. Una misura *spot* del Governo che ha operato in maniera sistematica per restringere al minimo la platea dei beneficiari, introducendo per molti un vero e proprio percorso ad ostacoli. Sulla beffa della carta acquisti come Gruppo abbiamo depositato una interpellanza e speriamo che il Governo voglia rispondere in tempi brevi. Come dicevo all'inizio, una misura inadeguata. Il nostro Gruppo già nel dibattito alla Camera, e ancora nelle Commissioni competenti, ha chiesto misure straordinarie all'altezza della straordinarietà della situazione. Una manovra dì un punto di 16 miliardi di euro per cercare di invertire la rotta, per un piano straordinario e universalistico per gli ammortizzatori sociali, per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Una misura in ritardo. Solo nei prossimi giorni si aprirà a Palazzo Chigi un tavolo di confronto sul settore dell'auto. Siamo già in ritardo, negli Stati Uniti e nei maggiori Paesi europei hanno già adottato o stanno in via di definizione pacchetti di misure consistenti per sostenere questo settore, settore che è la principale vittima della crisi internazionale e che è già sostanzialmente fermo da almeno un mese. Settore strategico per l'industria del nostro Paese che coinvolge, oltre ai propri addetti, centinaia di migliaia di lavoratori dell'indotto. E siamo ancora in attesa dell'apertura del tavolo di confronto, cosa aspettate? Cosa altro deve succedere? Il Mezzogiorno è sostanzialmente abbandonato a se stesso e vede decurtati gli stanziamenti per gli investimernti, così come gli enti locali che rischiano di essere soffocati da patti di stabilità interni che impediscono di programmare investimenti diretti e capaci di promuovere misure emergenziali di carattere sociale e per spese in conto capitale. Una manovra incerta: dagli inviti all'ottimismo del *Premier* alla cupezza del Ministro dell'economia e delle finanze, non vi è traccia di un'idea di come il nostro Paese possa uscire da questa situazione. Non c'è traccia di un'idea di politica industriale, non me ne voglia il ministro Sacconi, ma io sono tra quelli che pensa che in questo momento ce ne sia un gran bisogno, anche a rischio di essere etichettato come esponente di una sinistra vecchia e radicale. Non c'è un'idea unificante del Paese. Non si cerca il confronto con le forze d'opposizione, ma anzi, si lavora per dividere, a partire dalla frattura tra le parti sociali. Di ben altro si avrebbe bisogno: dovremmo ripartire dallo spirito del 1993. Il nostro Paese ha fortunatamente in sé una grande forza, quella che ci portò a superare la crisi finanziaria ed a portare il Paese nell'euro. L'ex presidente Ciampi, in una recente intervista, ha avuto modo di ripercorrere le vicende relative all'accordo del 1993, quando ha ricordato, che anche se in una fase diversa, un'intesa senza il maggiore sindacato, la CGIL, sarebbe stata semplicemente impensabile: «Ai miei tempi io» questo ha avuto modo di dire l'ex Presidente - «senza una componente della trattativa non sarei andato avanti». Lo spirito doveva essere quello di una concertazione tra tutte le parti sociali, non tra alcune sì ed altre no, a meno che non si voglia una rivincita sulla CGIL, una rivincita sul 2002, una rivincita sulla lotta per l'articolo 18. Ma di questo il Paese non ne ha bisogno. Temo che, a causa vostra, il Paese pagherà per questa crisi.

interveniamo in discussione generale su questo decreto anticrisi pur sapendo che ci sarà poco da modificare in questa sede; sappiamo però che nel corso dell'anno ci saranno altre occasioni importanti di intervento di politica economica. La situazione è abbastanza chiara sotto questo aspetto. La crisi evolve e, come si evolve la crisi, si evolvono le risposte dei differenti Governi. In estrema sintesi, che cosa andremo a sottolineare? Da un lato, quanto già va bene in questo decreto, dall'altro, quanto avremmo voluto inserire in più e di nuovo e, infine, una considerazione di carattere generale sulla situazione economica e sugli sviluppi che dovrà avere l'intervento di politica economica, che ci auguriamo ci coinvolga tutti in un confronto sereno e costruttivo. Di buono c'è parecchio in questo decreto. Partiamo dai pacchetti relativi alle imprese. Vi è anzitutto la revisione congiunturale degli studi di settore, aspetto fondamentale voluto dalla Lega Nord, che però vogliamo si sostanzi in tempi rapidi in risposte concrete agli imprenditori che stanno aspettando per capire cosa accadrà davvero agli studi di settori. Poi c'è il fondamentale emendamento - voluto dalla Lega alla Camera - salva Malpensa sulla liberalizzazione delle rotte, che conosciamo benissimo. Vi è quindi la questione dei rimborsi (finalmente un po' di rimborsi IVA, in particolare per le auto aziendali); c'è l'IVA per cassa per le aziende più piccole, la detassazione dei contratti di produttività, innovazione, efficienza organizzativa; la deduzione fino al 10 per cento di una quota dell'IRAP dall'IRES;

Casera a prendere nota di questa interpretazione autentica da dare all'articolo 30, in modo che sia chiaro che questo non è un termine «fino a», ma il termine di partenza per l'intervento sui confidi. Vi è inoltre l'eliminazione della commissione di massimo scoperto

primariamente sul Patto di stabilità degli enti locali, con una richiesta molto semplice: consentire gli investimenti ai Comuni virtuosi. E al riguardo avevamo previsto anche tre paletti per identificare tali Comuni: quelli che negli ultimi tre anni hanno rispettato il Patto di stabilità; quelli che non hanno l'addizionale IRPEF a livello massimo (altrimenti sono capaci tutti, perché basta aumentare le tasse) e, infine, quelli che hanno una media di personale inferiore alla media nazionale per fascia dimensionale.

In queste Aule abbiamo sentito per anni che lo studio di settore è una semplice statistica e non è una *minimum* *tax*; allora, è bene che sia una presunzione semplice, altrimenti è una presa in giro. rimettere gli ammortamenti anticipati e la deducibilità degli interessi passivi perché noi ci ricordiamo il male che ha fatto ai bilanci delle piccole e medie imprese quell'intervento a gamba tesa di Visco e Padoa-Schioppa. Questi sono due interventi molto importanti che danno davvero fiato alle imprese e, in particolare, a quelle che

un intervento senza un tetto. Ebbene, anziché mettere un tetto e limitare, si poteva agire molto meglio sulla base dei criteri tecnici, dando,

Passiamo - e mi accingo a concludere - a considerazioni di carattere più generale: dove si inserisce questo decreto cosiddetto anticrisi? Innanzitutto é stato giustamente rilevato dal relatore che

dimenticando quello che di più importante abbiamo fatto: anticipare i saldi finanziari a luglio e, quindi, stabilizzare l'economia del Paese per i tre anni futuri. Questo è quello che consente ed ha consentito al nostro Paese di affrontare serenamente questa crisi che è montata nel tempo.

del *rating* con pesantissimi effetti sul costo del servizio del debito. Fortunatamente, grazie alla prudente azione in politica economica mantenuta finora, noi non abbiamo avuto questo effetto. Purtroppo, pur a parità di *rating*, abbiamo uno *spread* che, come diceva giustamente il professor Baldassarri in precedenza, si mantiene eccessivamente elevato. Su ciò dobbiamo ancora agire per dare un segnale di chiarezza ai mercati.

Ecco, quindi una piccola rivincita del nostro modello, legato al sistema di piccole e medie imprese, al sistema di credito popolare cooperativo che sta dietro, al fatto che fortunatamente i nostri vecchi ci hanno insegnato anche a mettere da parte un po' di quattrini. Abbiamo dunque una propensione al risparmio tipicamente più elevata, che però, purtroppo in dieci anni si è ridotta di dieci punti. Quindi, qui dobbiamo intervenire, perché a furia di incentivare sempre un certo particolare mondo di grandi banche con un eccessivo accesso al credito al consumo, abbiamo un eccessivo accesso al credito al consumo, abbiamo messo sul lastrico parecchie famiglie. A volte, come si dice dalle mie parti, è meglio diventare rossi prima, che bianchi dopo. Se le banche, a suo tempo, avessero fatto un buon lavoro, affidando solamente chi ne aveva la possibilità

meglio. Abbiamo un'enorme opportunità; paradossalmente il fatto di avere una spesa pubblica così grande e fuori controllo ci dà un'enorme possibilità. Infatti, 780 miliardi di spesa pubblica sono una follia: per cento del PIL e del fatturato Italia. Solo il 5 per cento di taglio di una così enorme spesa pubblica fuori controllo ci dà 40 miliardi di euro all'anno,

Signora Presidente, come hanno rilevato molti colleghi, stiamo discutendo di un provvedimento che si colloca in un quadro congiunturale significativamente peggiorato rispetto al momento in cui il Governo lo adottò il 29 novembre scorso. Già questo ci indica la sostanziale irrilevanza delle misure previste dal decreto-legge in discussione e richiede di porsi nell'ottica di ripensare complessivamente la strategia degli interventi necessari a fronteggiare la pesante tendenza recessiva in atto. Nonostante le sollecitazioni e le proposte che abbiamo inutilmente avanzato da luglio, il Governo non ha sin qui messo in atto alcuna misura per una politica fiscale espansiva. Addirittura il cosiddetto decreto anticrisi di cui ci occupiamo attua una contrazione fiscale. Emblematiche sono, al riguardo, la rinuncia al meccanismo automatico per le norme sulle detrazioni a favore del risparmio energetico o per il sostegno alla ricerca, insieme con la limitata implementazione dei fondi ai consorzi fidi per le piccole e medie imprese. Allo stesso tempo, non si può però affermare che in Italia vi sia stata una politica fiscale davvero rigorosa. Sono state introdotte una serie di nuove imposte, come la cosiddetta *Robin tax*, che hanno un gettito molto aleatorio. Dopo la discutibile e poco rilevante operazione della *social card*, sono stati varati, con tale decreto-legge, un'infinità di microprovvedimenti (dal *bonus* famiglia all'intervento sui mutui, dalla detassazione dei premi di produttività alla deduzione dall'IRES di una quota IRAP e alla detassazione dei microprogetti di arredo urbano) di scarsa o modesta efficacia pratica, anziché concentrare gli interventi su alcune misure davvero prioritarie, nel senso ad esempio indicato dalle nostre proposte per una manovra aggiuntiva.

non serve a migliorare i conti pubblici e neanche a migliorare l'economia durante e, soprattutto, dopo la crisi. Dopo l'anticipo nella definizione dei cardini della manovra di politica economica dell'estate scorsa, il Governo si è ingessato; pur a fronte degli sconvolgimenti intervenuti, persiste in una colpevole inerzia. Nel frattempo, Germania, Regno Unito, Spagna e Francia hanno già adottato vari e consistenti pacchetti di misure, comprensive di rilevanti azioni di stimolo fiscale: siamo così l'unico grande Paese europeo a rimanere fermo di fronte a una grande recessione. È un atteggiamento che rischia di lasciarci più esposti e indeboliti, e per un tempo molto lungo, anche quando la tempesta si sarà calmata. In questo dibattito noi ribadiamo con forza che non c'è davvero più tempo da perdere: per aiutare imprese, lavoratori e famiglie in difficoltà, ma anche per rassicurare i mercati occorrono trasparenza e chiare scelte di politica economica contro la recessione. Rimanere in mezzo al guado, attestati sulla sponda di un rigorismo tignoso, come quello del Ministro dell'economia, in un singolare isolamento rispetto alle scelte di tutti gli altri Paesi europei, pur consapevoli dei margini margini ristretti entro i quali possiamo operare, è la peggiore soluzione possibile perché i conti si deteriorano senza migliorare le prospettive dell'economia. I dati sono lì a confermarlo:

Va sottolineato che in queste stime si prescinde da ulteriori effetti peggiorativi dipendenti dall'indebolimento delle misure antievasione, già adottate con il decreto di luglio e a seguito dell'applicazione delle disposizioni previste anche in questo decreto anticrisi. Del resto, ed eravamo stati facili profeti, la lotta all'evasione fiscale, che pure a parole è un obiettivo dichiarato dal Governo, sta andando chiaramente male. scontare il fatto che il Governo non ha presentato al Parlamento il *report* sulla lotta alla evasione ed elusione previsto dalla finanziaria 2007 a cui da settembre scorso era tenuto, a causa del peggioramento della *tax compliance* e dell'aumento dell'evasione fiscale, si può stimare che nel 2008 siano stati persi circa 6-8 miliardi di euro di entrate rispetto a quelle prima recuperate al fisco. La cosa non deve stupire: si raccoglie quanto seminato. È dal primo decreto di finanza pubblica di maggio a questo di cui discutiamo che denunciamo, inascoltati e mal sopportati, nella generale disattenzione degli organi di informazione, che in soli sei mesi sono state smantellate le principali misure antievasione approvate precedentemente dal Parlamento e che si è ridotto drasticamente il sistema sanzionatorio. Questo è avvenuto già con l'introduzione dell'adesione alle verifiche fiscali con sconto delle sanzioni, disposte dal decreto n. la misura estremamente bassa della sanzione è un premio, e incentiva di fatto i comportamenti scorretti, oltre a risultare paradossalmente più conveniente di quella dovuta dal contribuente che, mediante ravvedimento operoso, cioè spontaneamente e senza intervento dell'amministrazione finanziaria, corregga la propria dichiarazione fiscale. In questo decreto sono stati introdotti ulteriori interventi, che in parte correggono quella distorsione per fortuna, ma soprattutto configurano nuove opportunità a favore dei contribuenti scorretti. queste norme sono un'evidente conferma del lassismo fiscale che caratterizza l'azione del Governo. L'obiettivo potrebbe sembrare quello di accelerare la riscossione delle imposte accertate. In realtà, anche a voler ammettere che queste norme possano determinare qualche incremento di gettito nelle riscossioni da accertamento (il che è tutto da dimostrare), è certo che esse determineranno maggiore evasione in termini di adempimento spontaneo, sul quale si regge, come è noto, la gran parte del gettito tributario. D'altra parte, è dimostrato che, ferma restando la numerosità dei controlli che l'amministrazione è in grado di effettuare, l'evasione tende ad essere più elevata quanto più basse sono le sanzioni. Dunque è un modo veramente strano di condurre la lotta all'evasione. Così si rinuncia ad incidere sull'unico terreno che potrebbe recuperare risorse ingenti, introdurre fattori di trasparenza, innovazione e competitività nell'economia, tenere insieme e far interagire modernità e civismo. In realtà, si fa tutto il contrario di ciò che sarebbe davvero necessario, perché il rapporto fisco-contribuente in Italia soffre di insostenibile sperequazione: enorme evasione fiscale, peso eccessivo delle imposte, pessima e iniqua distribuzione del carico fiscale.

Si prevede che, per tenere conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell'economia, questi possano essere rivisitati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche dopo la data del 31 marzo. Insomma, lo dico al senatore Garavaglia che ne ha parlato, dopo tante promesse e retorica, la montagna ha partorito un topolino: parole, un lenimento quasi fosse la coperta di Linus. Occorre invece prendere atto che la crisi colpisce tutti i settori dell'economia e che per l'anno 2008 i rischi di una eventuale non congruità per i contribuenti con partita IVA sono elevati. Dunque, almeno sugli studi di settore per l'anno 2008, dovrebbe essere invertito l'onere della prova, come prevede peraltro la mozione approvata dal Senato nel luglio 2007, e come aveva disposto l'Agenzia delle entrate, con propria circolare rispettosa degli indirizzi del Parlamento. Ma l'ineffabile ministro Tremonti ha detto di no, perché un conto sono le parole di propaganda, ben altra cosa è quando si prendono le decisioni vere. Anche in questo caso, un'ulteriore significativa dimostrazione della distanza abissale tra enunciazioni e comportamenti, in cui si distingue questo Governo, e la conferma che bisogna la più presto cambiare stile, comportamenti e, soprattutto, le scelte. legge n. 1315** Signora Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,

non può prescindere da uno sguardo attento al settore primario, che rappresenta una delle vocazioni più radicate nel Paese. Da un complesso di provvedimenti che dovrebbe incentivare il lavoro, l'occupazione, l'impresa e dico testualmente - «ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», sarebbe legittimo, oltre che verosimile, attendersi anche misure finalizzate al sostegno ed al rilancio dell'agricoltura;

anche attraverso il Governo ombra, all'interno del quale sono incaricato di seguire questi temi, aveva segnalato da subito, e cioè sin dall'inizio della legislatura, la sofferenza del comparto, mentre ai suoi danni, con altrettanta tempestività, il Governo operava vistosi tagli. Successivamente, quando è esplosa la crisi economica, abbiamo ribadito la necessità di interventi a favore dell'agricoltura mediante i provvedimenti che via via si susseguivano. Sostanzialmente abbiamo sempre registrato una sorta di refrattarietà da parte del Governo, quasi a voler negare l'evidenza della criticità che interessava e interessa il settore. L'unica eccezione in questo primo scorcio di legislatura si è verificata in occasione della conversione in legge del decreto-legge sulla competitività nel settore agroalimentare: non ripeterò quanto già detto in altre circostanze. Mi limito in sintesi a ricordare che in prima lettura al Senato il Gruppo PD presentò significativi emendamenti che la Commissione agricoltura licenziò all'unanimità, Aula dai colleghi della maggioranza. Una parte considerevole di quegli emendamenti fu poi ripresentata alla Camera dei deputati dal PD, finalmente incontrando l'assenso del Governo. E dunque, tornando al Senato, il decreto ricevette il definitivo via libera. Solo così

e di una effettiva volontà di rilancio competitivo del settore, valorizzando le tante eccellenze del *made* *in Italy* e favorendo una più adeguata attività di promozione. Anzi, c'è di più:

qualche modesta attenzione, capita che alla prima occasione successiva il risultato conseguito venga ridimensionato, quasi sempre a causa della riduzione dell'originario affidamento finanziario. Qui siamo all'inverosimile: la *Gazzetta Ufficiale*, il 30 dicembre 2008, ha pubblicato la conversione in legge del decreto sulla competitività nel settore agroalimentare: cioè quanto i due rami del Parlamento aveva pochi giorni prima approvato. Il 31 dicembre (il giorno dopo!) con il cosiddetto decreto milleproroghe il Ministro dell'economia vi ha apportato modifiche che colpiscono naturalmente l'agricoltura e la pesca. Mi riferisco alla copertura finanziaria - già non molto significativa rispetto al reale fabbisogno - del credito d'imposta per l'internazionalizzazione delle imprese agricole, alla questione relativa al canone ricognitorio per le cooperative ittiche, ed ancora all'interpretazione autentica del contenzioso INPS, negando, così, i benefici alle piccole cooperative agricole. Sono perciò fondate e forti la delusione e la preoccupazione degli imprenditori del settore, molti dei quali vedono a rischio la tenuta delle proprie aziende e il mantenimento dei livelli occupazionali. Il dato di fronte al quale ci troviamo non è certo incoraggiante: nel terzo trimestre del 2008 si è verificato rispetto al precedente un calo del 3 per cento del valore aggiunto in agricoltura, anche se il dato tendenziale (più 4,5 per cento) resta positivo.

Il decreto anticrisi interviene su una sola questione che ha afferenza con le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dunque delle Commissioni corrispondenti del Senato e della Camera: le le disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (cosiddetto PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento dell'UNIRE e del CONI. Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'UNIRE è determinata in 150 milioni.

allo scopo di incrementare il montepremi e le provvidenze per l'allevamento dei cavalli, e in parte al CONI e allo stesso UNIRE in funzione del loro risanamento finanziario e del riassetto dei relativi settori. Vengono escluse le ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE. Concludendo, naturalmente il Gruppo del PD riproporrà gli emendamenti relativi al Piano irriguo nazionale, all'estensione del credito di imposta nel settore agroalimentare, al Fondo di solidarietà nazionale, alle incentivazioni per l'imprenditorialità femminile e giovanile, al fondo per il *made in Italy.* II Gruppo del PD, inoltre, esprime preoccupazione per la superficialità con cui il Governo tratta un tema così centrale nell'economia nazionale come l'agricoltura e francamente - spiace dirlo - rileva quanto sia marginale il ruolo del Ministero competente, che non riesce ad affermare il proprio peso all'interno dell'Esecutivo, a reclamare il rispetto dei diritti del settore primario e ad ottenere riconoscimenti dignitosi

disegno di legge n. 1315** Fin dai primi atti di questo Governo ci siamo dovuti abituare a provvedimenti onnicomprensivi che trattano di tutto, dove le singole questioni sono prese e riprese più volte, in testi diversi ed in occasioni diverse. Tutta la manovra finanziaria è stata realizzata così, e così si presenta anche questo decreto-legge. Non sottolineo quest'aspetto per un astratto bisogno di metodologie normative catalogatorie, ma per sottolineare un metodo di lavoro confuso, tutt'altro che trasparente e spesso poco chiaro. Allora è inutile decantare il fatto che si siano eliminate, per semplificare, 3.000 leggi e poi tutto in realtà, giorno dopo giorno, provvedimento dopo provvedimento, risulti più arzigogolato e confuso di prima. Ma soprattutto è difficile scorgere con chiarezza quali sono le priorità e se esiste una linea unificante di iniziative a contrasto della crisi, intorno alle quali potersi confrontare utilmente e quindi mobilitare tutte le risorse di questo Paese. Invece il Paese è stato lasciato solo di fronte ad una delle crisi più gravi che si siano affrontate nella storia moderna. I pensionati, i giovani, i lavoratori, gli imprenditori, i professionisti, le famiglie dovranno contare solo sulle proprie forze con il rischio di rimanere chiusi nei propri interessi e nei bisogni più prossimi. Gli eventi degli ultimi mesi, i dibattiti, le scelte che altri Paesi stanno facendo in questi giorni ci dicono che senza un impegno corale e condiviso sarà impossibile uscire da questa crisi più forti, più civili e più competitivi. Nell'articolo 2-*ter*, dove si tratta dell'utilizzo del risparmio degli enti locali, si scorge un approccio metodologico interessante sulla questione del vincolo di stabilità che, se approfondito adeguatamente, avrebbe permesso forse di individuare e sperimentare, nello specifico della crisi, percorsi virtuosi d'intervento collocabili oltre l'astratta, rigida difesa della tutela del Patto di stabilità e senza sollecitare eccessi opposti. Ma la strada scelta dal Governo non è stata questa e il decreto in esame, per il suo carattere di sostanziale neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica per il prossimo triennio, si muove in direzione opposta agli interventi che si stanno realizzando negli altri Paesi europei. Ci avviamo dunque a discutere di un decreto che contiene per la gran parte interventi a costo zero, mentre la crisi dilaga e tocca ormai la maggioranza della società italiana, dai piccoli e medi imprenditori ai lavoratori licenziati o in cassa integrazione, ai precari (che sono i primi a perdere il posto di lavoro), alle famiglie e ai pensionati. 30 decreti-legge e 10 voti di fiducia (che spero non diventino undici domani) non sono stati sufficienti a comporre una vera manovra di bilancio, in grado di spostare risorse reali verso l'economia, il lavoro e le famiglie. La denuncia dell'opposizione riguarda anche il rischio concreto che la manovra economica, permanentemente in corso da otto mesi, non sia ancora finita e che ulteriori provvedimenti dovranno essere emanati per finanziare gli ammortizzatori sociali ed altre emergenze. La maggioranza ha sostenuto alla Camera che l'opposizione fa del pericoloso pessimismo, ma i dati dicono che la produzione industriale a novembre è calata del 12,7 le piccole e medie imprese faticano ad avere linee di credito; migliaia di esercizi commerciali hanno chiuso; crescono in modo esponenziale le ore di cassa integrazione; i consumi si riducono. Il Governo obietta che la crisi non si può attribuire alla sua responsabilità, alla responsabilità del Governo è da attribuire l'assoluta mancanza di un'idea per trascinare il Paese fuori dalla crisi. Signora Presidente, consegnerò il testo integrale del mio intervento, ma una cosa mi consenta di dirla ancora. In questo decreto non si parla di turismo. Per questo settore, che è uno dei pochi

potuti utilizzare in questo provvedimento.

Mi permetto di rivolgerle un invito: domani cerchi di intervenire anche lei su questo argomento, rammentando a noi tutti parlamentari di essere per primi più ossequiosi del Parlamento, perché tutte le discussioni generali sui provvedimenti vedono presente meno di una trentina di parlamentari. Questo è segno di poca dignità per il Parlamento italiano, soprattutto per alcuni parlamentari - e mi riferisco, ad esempio, al Vice presidente del Gruppo del PD, senatore Zanda, che spesso fa interventi

ad approvare questo provvedimento e il Parlamento è stato obbligato ad integrarlo, per quanto ha potuto, alla Camera dei deputati, e noi al Senato abbiamo ovviamente una funzione meramente notarile dato che dopodomani il decreto, se non fosse approvato, andrebbe a scadere. scadere. Vorrei richiamare la sua attenzione su un qualcosa che non è stato fatto e che poteva essere fatto micro e piccola industria, signor Sottosegretario. Lei sa benissimo che i limiti del capitalismo italiano sono proprio il nanismo delle imprese e la loro modesta patrimonializzazione. Ebbene, c'erano due provvedimenti che potevano essere assunti e che non si sono concretizzati; per uno, in verità, parzialmente si è fatto qualcosa, ma avremo modo di vedere in futuro che è del tutto insufficiente.

ma nella misura di una tassazione del 7 per cento che di sicuro non attrarrà l'interesse di alcuna azienda. Pertanto, le anticipo che, ad una interpellanza già presentata, su cui attendo ancora risposta su di un altro argomento che di qui a poco le richiamerò all'attenzione,

del 7 per cento è del tutto impossibile che in un momento di tale crisi, soprattutto di liquidità, le imprese possano usufruire di questa attenzione del Governo. L'altra misura che non è stata proprio affrontata è quella che prevede di facilitare gli accorpamenti delle micro e piccole imprese. A suo tempo, per il mondo bancario furono predisposte delle agevolazioni; in questo provvedimento non c'è nulla per favorire la crescita delle piccole imprese italiane. Quando ricordavo il titolo pomposo del disegno di legge che nasce da una crisi mondiale,

di interventi per il mondo automobilistico. Sarebbe il caso di capire che c'è un tessuto produttivo del Paese che non riesce ad avere alcuna attenzione. Signor Sottosegretario, parlo da imprenditore: abbiamo ascoltato in Commissione industria il presidente della piccola industria, il quale ha fatto riferimento (lo ricordo ai commissari,

Credo che bisognerà tornare su questo, anche perché la crisi di cui tanto si parla e che in Italia subiamo ha delle origini

di conversione del decreto-legge n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa, non può non considerare la gravità della crisi economica in atto. Come è stato ricordato nel corso di questo dibattito, si tratta di una crisi finanziaria internazionale che riguarda sempre più l'economia reale, come testimoniano i dati diffusi

dell'Unione europea una recessione profonda e prolungata, con un aumento della disoccupazione di circa tre milioni e mezzo di unità. Per l'Italia si prevede una riduzione del prodotto interno lordo del 2 per cento e un aumento, secondo i dati di Confindustria, della disoccupazione di almeno 600.000 unità. Dovremo quindi affrontare una recessione profonda, che è già in atto e che si riflette con un forte calo degli investimenti, delle esportazioni e dei consumi, calo che ha moltiplicato in questi ultimi mesi il ricorso alla cassa integrazione. Di fronte a un quadro economico di tale natura e gravità, il Governo in carica, dopo le misure depressive varate nei mesi scorsi con la manovra triennale e confermate nell'ultima legge finanziaria, oggi propone, con il disegno di legge in discussione, interventi *una tantum* e misure insufficienti e inaccettabili.

come peraltro hanno sostenuto nei giorni scorsi sia il Presidente del Consiglio che il Ministro dell'economia. europei, come la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, la Spagna, stanziano risorse ingenti per cercare di contenere questa drammatica emergenza, il Governo italiano minimizza e fa delle battute. Noi del Partito Democratico pensiamo invece che per fronteggiare questa drammatica situazione sia indispensabile prevedere una manovra aggiuntiva pari almeno è parlato di 16 miliardi - per affrontare soprattutto due emergenze: la necessità di attuare al più presto una riforma organica degli ammortizzatori sociali e un un innalzamento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, autonomo e da pensione. Se vogliamo davvero perseguire tutto questo, perseguire tutto questo, si richiedono un confronto franco e aperto con l'opposizione ed una forte coesione sociale. Il Governo invece, ancora una volta, ha scelto la strada del voto di fiducia, che probabilmente

esame, palesemente carente nel fronteggiare la grave crisi economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese in maniera preoccupante. Le ricette economiche sinora proposte dal Governo non sono state né immediate, né adeguate ad affrontare alcun aspetto strutturale dell'attuale crisi per difendere i salari, i posti di lavoro e per rilanciare i consumi. L'ammontare degli interventi contenuti nel decreto anticrisi ha un valore di 4,9 miliardi di euro, una cifra modesta anche rispetto agli interventi messi in atto da altri Paesi europei che hanno stanziato ingenti risorse a sostegno dei settori strategici per il loro sviluppo economico ed ambientale, prevedendo una riduzione della pressione fiscale a vantaggio delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie. modesta anche rispetto ai provvedimenti attuati dalle Regioni in favore delle famiglie e delle imprese per un valore complessivo superiore ai 2,5 miliardi d'euro, a cui si aggiungono i Fondi europei e quelli destinati a confluire negli armonizzatori sociali a declinazione territoriale. Si deve dare atto che, mentre le Regioni sono intervenute sul terreno più importante su cui si gioca la partita anticrisi, cioè il sostegno alle imprese che da solo assorbe il 60-65 per cento dell'impegno finanziario finora messo a bilancio dalle medesime, lo Stato, pur avendo maggiori risorse, non è intervenuto con mezzi e strumenti consistenti. Non possiamo non rilevare poi come il Governo abbia ancora una volta sottovalutato la crisi finanziaria e non considerato immediatamente che la stessa avrebbe travolto l'economia con conseguenze e danni gravissimi per la produzione. In merito al provvedimento in esame desidero evidenziare alcune problematiche. L'articolo 9 prevede, solo per l'anno 2009 e nei termini ivi normati, tempi di pagamento ridotti da parte della pubblica amministrazione. Ritengo che la certezza e il rispetto dei tempi di pagamento fissati siano irrinunciabili per la sopravvivenza delle aziende che operano con l'amministrazione pubblica e devono sussistere sempre senza alcuna condizione e/o limitazione. Le risorse destinate poi al *bonus* straordinario, *una tantum,* previste dall'articolo 1 per famiglie, lavoratori, pensionati e la non autosufficienza sono largamente insufficienti e non spettano indistintamente a tutte le persone che si trovano in una determinata condizione, ma sono attribuite unicamente rispettando l'ordine cronologico della presentazione delle domande, con la grave conseguenza di escludere una considerevole quantità di persone. I criteri previsti per usufruire dei benefici sono molto restrittivi e i requisiti richiesti si presentano contradditori: le famiglie titolari di redditi per immobili in affitto o titolari di piccoli terreni con redditi di modestissima entità, per esempio,

Negli articoli 18 e 19 sono previsti interventi sugli armonizzatori sociali e i fondi stanziati per finanziare gli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro di disoccupazione risultano essere inadeguati e insufficienti rispetto alla platea di persone alle quali si riferiscono i benefici. Forse sarebbe stato meglio adottare una riforma più organica. Basti pensare che in questi giorni nella mia piccola realtà altre due fabbriche con oltre 200 dipendenti chiuderanno i battenti.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento probabilmente più di altri costituisce la rappresentazione quasi plastica della inconsistenza di questo Governo. Un Governo mediatico, la cui azione è prevalentemente, se non esclusivamente, improntata alla sola efficacia mediatica. Un Governo quindi molto abile ad occupare tutti gli spazi televisivi possibili e a veicolare messaggi *spot* ad effetto, ma che dietro la propria apparenza dimostra davvero poco o niente. Non credo che si possano occultare alla lunga gli effetti di questa crisi, pensando di ammorbare o narcotizzare l'opinione pubblica. Ci troviamo oggi probabilmente solo all'inizio di una crisi che, per quanto sia ancora non definibile con certezza nelle dimensioni e nella durata, avvertiamo comunque essere significativa ed intensa. Una crisi che chiama direttamente in causa l'intervento e l'azione pubblica dei Governi nazionali, con uno *stock* di misure importanti sia qualitativamente che quantitativamente: dalla predisposizione di ammortizzatori sociali - come è stato ricordato - soprattutto a chi non ne dispone ad interventi di sostegno e ricapitalizzazione a significativi comparti della produzione e del credito. crisi, i Governi dei principali Paesi europei seguono l'imponente sforzo statunitense, assecondandolo con interventi straordinari quantificabili da tre a cinque punti percentuali del proprio prodotto interno lordo.

che probabilmente qualcuno glielo deve dire al manovratore che non vuole essere disturbato che la crisi è reale, che non è una crisi virtuale,

Voglio evidenziare che il problema da oggi non è probabilmente solo di segno, cioè vi è la necessità non solo di una manovra moderatamente di intonazione espansiva, ma anche, probabilmente da domani, di un coordinamento con le politiche economiche comunitarie. comunitarie. Non credo che possa risultare agevole né a Berlusconi né tanto meno a Tremonti cavarsela in quella sede con un piatto di ottimismo, reclamato da noi, nel nostro Paese, nei confronti dell'opinione pubblica

che oggi approda in quest'Aula con una probabile conclusione blindata, in realtà sono per 3 miliardi il rifinanziamento in ben 15 anni della legge obiettivo e per un miliardo e mezzo le risorse assegnate a Ferrovie dello Stato sul fondo investimenti e per la stipula dei contratti regionali che il Governo aveva dimenticato di inserire in finanziaria. risorse sono esattamente in linea con gli stanziamenti storici del settore, pari cioè a quelli che nei precedenti anni aveva stanziato il Governo Prodi. Per il resto, se si eccettua il rifinanziamento dell'IMA, cioè dell'indennità mancato avviamento per i lavoratori portuali, pari a 12 milioni (è una piccola cifra, che però risolve un problema importante), sono soltanto norme, forse utili, ma solo se a queste seguiranno le risorse. mi rivolgo ai pochi colleghi della maggioranza ancora presenti - che presto o tardi questo atteggiamento, che giudico spavaldo e noncurante dei problemi reali, rischierà di trasformarsi in un *boomerang* nei cittadini temo davvero in grado di travolgere tutto. Vi potrà sembrare paradossale, ma siamo preoccupati anche dall'opposizione per la tenuta delle istituzioni democratiche. Noi riteniamo che le crisi costituiscano, invece, anche una inevitabile occasione di trasformazione e che, per quanto dolorose (e questa indubbiamente già lo è), possano rappresentare un'opportunità per rafforzare e consolidare gli *asset* positivi di un sistema. Sicuramente questa sarà una crisi che non ci vedrà uscire nello stesso modo in cui ci siamo entrati. È una crisi economica che ha prodotto implicazioni finanziarie inedite, ma non dimentichiamo che, in primo luogo, è una crisi etica, fatta di comportamenti, scelte e azioni conseguenti, individuali e collettive, assolutamente intollerabili. Il capitalismo è ben lungi dalla sua fine, ma la necessità di una sua profonda rivisitazione nelle regole mi sembra davvero ormai questione all'ordine del giorno. L'assenza e la distanza da queste riflessioni dell'attuale Governo lo connota più come un Governo balneare anziché di salute pubblica, di cui vi sarebbe la necessità per i problemi davvero enormi che sono in gioco.

su un provvedimento definito in maniera sostanziale dall'altro ramo del Parlamento, che al testo originariamente proposto dal Governo ha apportato significativi miglioramenti. Vorrei brevemente citare, ad esempio, il ripristino di quel famoso *ecobonus*, che dall'opposizione ci viene contestato e che invece abbiamo salvaguardato, oppure l'introduzione di modifiche agli ammortizzatori sociali (che noi consideriamo importantissimi), o le misure in materia di accertamento fiscale. Il Senato negli ultimi mesi è stato molto impegnato su diversi fronti, alcuni molto importanti, direi importantissimi, come ha ricordato in precedenza il relatore Conti (solo la settimana scorsa è stato licenziato il notevole testo sul federalismo fiscale) e questa densa attività ha costretto questa Camera ad una ridotta seppur approfondita analisi in sede di Commissioni riunite del decreto in esame. Spero che quest'Aula voglia esprimere il proprio assenso ad un provvedimento importante - non a caso è stato dichiarato collegato alla legge finanziaria approvata nel dicembre scorso - sia nella struttura e nel contenuto che nelle finalità più generali. Un provvedimento che rientra nel quadro più ampio della politica economica che il Governo ha messo in atto dall'inizio del suo mandato e che deve tener conto della peculiare struttura della finanza pubblica italiana. Guai se ci dimenticassimo di questo! Un intervento di oltre 6 miliardi di euro, che si inserisce nel contesto di interventi comunitari volti a fronteggiare la pesante crisi internazionale: il piano di ripresa economica deliberato in sede di Unione europea per 200 miliardi, di cui 170 derivanti dai bilanci nazionali e 30 dalle risorse della Unione europea e della Banca europea che prevedeva interventi tempestivi e temporanei, combinazioni di strumenti di reddito e di spesa. Il provvedimento in esame è, a nostro avviso, una risposta adeguata all'attuale momento, articolandosi su due grossi filoni di intervento: da un lato, l'azione su chi sta meno bene e chi è più sfortunato e quindi più esposto a questa fase economica, sulle fasce di reddito più deboli quindi, e, dall'altro, la stabilizzazione del sistema non lo dobbiamo dimenticare - ha travolto altri Paesi, mentre invece, in virtù dell'intervento del Governo italiano e di una storia e di una struttura diverse dalle banche italiane, è per noi è per noi motivo di maggiore e cauto ottimismo rispetto alla crisi che avanza. Il decreto, infatti, contiene misure che qualcuno legittimamente potrebbe giudicare insufficienti, ma che in realtà, non appaiono affatto Basti pensare, per esempio, al *bonus* per le famiglie (che ammonta solo per il 2009 a circa 2,5 miliardi di euro), all'integrazione del Fondo per l'occupazione (che assomma nel triennio risorse per oltre 800 milioni di euro), al contributo in conto interessi per i mutui (verso cui sono stati stanziati 300 milioni di euro per il 2009 e 20 milioni per sostenere l'accesso alle case in locazione).

e alla composizione delle famiglie utilizzati nell'articolo 1 del provvedimento aprono in qualche modo un spiraglio verso la possibile costruzione di una fiscalità orientata al nucleo familiare: quel famoso coefficiente familiare che in altri Paesi è già applicato ed ha dato ottimi risultati. Se è vero che il problema principale in questo momento è sostenere la domanda,

Così come non può essere sottovalutata l'azione concretamente intrapresa verso le imprese in materia di deducibilità dell'IRAP, ai fini dell'IRES e dell'IRPEF, con oltre 2,3 miliardi di euro nel triennio; misure che si accompagnano a quelle finalizzate al finanziamento, mediante il potenziamento della garanzia statale per i confidi, ovvero la sottoscrizione pubblica di obbligazioni, intervento quest'ultimo che appare garantire anche la necessaria stabilizzazione e l'adeguato rafforzamento dell'assetto patrimoniale delle nostre aziende di credito. Inoltre, non credo sia generosa la critica avanzata da alcuni colleghi dell'opposizione circa il presunto allentamento dei controlli sul rispetto dell'obbligazione tributaria e sulla lotta all'evasione. invece ricordare che il provvedimento reca misure specifiche in materia di accertamenti e riscossioni per importi assai rilevanti. Sul tema dell'evasione fiscale - lo voglio ricordare al senatore Barbolini - non accettiamo lezioni e non ci stancheremo mai di ricordare cosa sono stati due anni del Governo Prodi in termini di aumento della pressione fiscale. Il Governo Berlusconi lasciò la pressione fiscale al 41 per cento e questa fu aumentata dopo pochi mesi di Governo Prodi, dal primo decreto Visco-Bersani;

ci si chiede di diminuire la pressione fiscale in un momento di crisi difficilissima. Noi di certo lo faremo e continueremo a farlo (lo ha ricordato meglio di noi il presidente della Commissione finanze Baldassarri), ma ricordiamo soprattutto a questa opposizione che che quando lo si poteva fare non lo si è voluto fare, nonostante le nostre richieste e la preghiera che saliva dal Paese. Strozzate le aziende da una pressione fiscale così forte oggi pretendiamo che queste affrontino la crisi, soprattutto dal punto di vista finanziario,

Accennavo all'inizio dell'intervento che il provvedimento in esame è stato emanato con una particolare attenzione alla situazione della finanza pubblica, perché il tema della finanza pubblica è strettamente correlato con quello delle tasse, come dimostra la nostra storia. Il provvedimento presenta un limitato impatto correttivo - in senso migliorativo - sui saldi di riferimento (saldo netto da finanziare, indebitamento e fabbisogno) e non poteva essere Il nostro Paese, infatti, soffre del peso che comporta il terzo debito pubblico del mondo e i margini di intervento sono estremamente ridotti. Il Governo, quindi, ha giustamente ritenuto di non definire misure di politica economica in deficit, sebbene anche in Europa ci sia una generale propensione a giustificare l'attenuazione dei vincoli del Patto di stabilità;

In una situazione come la nostra un peggioramento dei saldi di finanza pubblica sarebbe insostenibile, come ha ricordato il presidente Baldassarri nel corso della discussione nelle Commissioni riunite in sede referente. Appare, quindi, quanto mai necessario rispettare la decisione di mettere in sicurezza i conti pubblici e mantenere questa linea, attuata inizialmente con la manovra estiva e consolidata con la più recente legge finanziaria.

dovuto fare i conti con una situazione di finanza pubblica devastante, generata e iniziata dal Governo Prodi e che noi siamo riusciti a fermare.

l'Unione europea potrebbe piombare in una recessione profonda e duratura, registrando un'ulteriore contrazione dell'economia e della disoccupazione. Questa affermazione scaturisce da un'analisi che non è frutto del catastrofismo dell'opposizione, ma è la disamina puntuale della situazione basata sulle previsioni fatte dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. analisi ha portato il presidente della Commissione Barroso e il presidente della Banca centrale europea Trichet a lanciare, ancora in questi giorni, un grido di allarme ai Governi nazionali perché si muovano tempestivamente, energicamente ed in modo coordinato nella definizione di interventi produttivi e strutturali, che affrontino l'emergenza ma costruiscano il futuro. È evidente che prendere atto della situazione e chiedere un'azione rapida e decisa per bloccare questa spirale negativa non è ritenuto da Barroso e da Trichet irresponsabile catastrofismo ma, viceversa, un obbligatorio segno di responsabilità e coraggio. Sappiamo che la situazione dell'Italia non è tra le migliori dell'Unione europea, tant'è che a fronte della previsione di crescita zero di molti Paesi la nostra sarà negativa; ma evidentemente questo Governo pensa che dichiarazioni ottimistiche, incitamenti alla fiducia e un lungo elenco di misurine da «Monopoli», siano sufficienti per un Paese che non ha un sistema di ammortizzatori sociali sufficiente né un dignitoso piano di rilancio dell'economia che, per esempio, preveda, a fronte di dati più negativi rispetto agli altri Paesi, un forte e deciso rilancio dell'occupazione femminile, valutato dalla Strategia di Lisbona come uno degli assi portanti della crescita economica. Brilla in questa situazione la pigrizia di questo Governo, che ritarda nel recepimento della direttiva di parità tra uomini e donne nel mercato del lavoro e si limita ad annunci allarmistici sull'innalzamento dell'età pensionabile delle donne senza prevedere un quadro di intervento sistemico che includa una normativa del lavoro delle donne, la parità salariale, incentivazioni fiscali, sostegno alla carriera professionale e alla conciliazione familiare e asili nido. A ben vedere, un dibattito serio sulla direttiva parità e sulla sentenza della Corte di giustizia europea in materia di pensioni delle donne nel pubblico impiego ci offrirebbe la possibilità di confermare che non si tratta tanto di innalzare l'età pensionabile delle donne, ma di mettere tutti, uomini e donne, sullo stesso piano in un quadro di flessibilità e con azioni positive per recuperare lo svantaggio delle donne. Questo chiede la sentenza, questo chiede l'ordinamento europeo. Per questo siamo pronte a dare il nostro sostegno in questa Aula. Stupiscono pertanto le intenzioni di quanti pensano di poter far cassa sulle spalle delle donne. Quello che non finisce di stupire è che i tre Fondi di sostegno all'occupazione femminile e giovanile varati dal precedente Governo sono stati asciugati dall'attuale Governo e convogliati in uno solo, che prevede 150 milioni di euro per il solo 2008, senza che peraltro sia mai stato fatto il decreto attuativo. Al danno si aggiunge la beffa! Stesso discorso vale per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, che il Governo vuole effettuare senza oneri per il bilancio nonostante l'Europa sia disponibile a flessibilizzare il Patto di stabilità. Dopo la scelta di togliere l'ICI anche ai più ricchi, dopo la vicenda Alitalia-Air France, si procede sulla strada dei tagli al cofinanziamento nazionale al Fondo sociale europeo erogato alle Regioni per far fronte alla formazione dei lavoratori. un'altra scelta non allineata alle misure di sostegno del reddito e di preparazione professionale che l'Unione europea prevede. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. Adesso ampiezza e profondità della crisi sono note e quindi stupisce come i partiti a forte connotazione popolare che stanno nella maggioranza possano continuare a guardare ad altro.

risposta infatti, anche se più o meno fastidiosa, ingombrante o problematica, ruota attorno al concetto di europeizzazione. Parlando perciò di politiche anticrisi non ci si può non riferire in primo luogo al programma di lavoro della Commissione per il 2009, dove sono individuate dettagliatamente le azioni da compiere nei quattro settori prioritari della Strategia di Lisbona. In questo senso la Commissione ha presentato relazioni individuali sui singoli Stati membri, comprendenti proposte di raccomandazioni, che vanno dall'occupazione alle tutele sociali, al sistema delle imprese, alle infrastrutture ed energia, alla ricerca ed innovazione. In altri Paesi tale quadro di riferimento ha determinato la nascita di un forte partenariato tra il pubblico ed il privato, come ad esempio nel settore automobilistico, a fronte però di innovazioni radicali, auto verdi, fabbriche del futuro, trasporto pubblico pulito. L'Europa mette quindi in campo tutti gli strumenti di cui dispone, invitando gli Stati membri a collaborare e coordinarsi con l'Unione per contribuire a una più vasta risposta globale. Tocca adesso agli Stati membri avvalersi dei punti di forza dell'Unione, nonché dei vantaggi di scala offerti dall'euro e dal più grande mercato unico del mondo. A tale proposito è bene ricordare che la maggior parte degli strumenti di politica economica, quelli necessari ad incentivare la domanda dei consumatori a breve termine, è in mano agli Stati membri; è bene altresì ricordare che interventi nazionali adeguatamente coordinati possono perseguire parallelamente scopi diversi ed attenuare le conseguenze della crisi, ma devono promuovere anche riforme rispondenti ai bisogni di lungo periodo per uscire più forti dalla crisi, definendo il giusto *mix* di misure tra consolidamento,

sotto il profilo sociale e sia sbagliato sotto il profilo dell'interesse generale. In generale, soprattutto in tempi di emergenza economica, il ruolo dell'opposizione e delle forze sociali è più che mai indispensabile. Colleghi, il confronto è utile, ma lo è prima, di un decreto-legge imposto con il voto di fiducia per problemi interni alla maggioranza, alla sua coesione e compattezza. rimaniamo aperti al confronto nell'interesse dell'Italia, aperti soprattutto nel discutere una manovra aggiuntiva di cui c'è urgente bisogno nel nostro Paese.

crisi la smettessimo di agitare le bandierine dei meriti o dei demeriti; credo che il nostro Paese abbia bisogno di un senso di grande responsabilità da parte di ognuno di noi. Pertanto eviterei di parlare di Prodi; anzi, è grazie a Prodi se oggi abbiamo i conti messi meglio di come meglio di come la precedente maggioranza li lasciò nel 2006; è sempre grazie a Prodi e a Ciampi se abbiamo l'euro. Ricordiamoci quanti rappresentanti centrodestra, che oggi sono al Governo, hanno criticato quel tipo di scelta. Oggi ci sono Paesi, decantati fino a pochi mesi fa, che vorrebbero entrare nell'euro perché sono nel mezzo di una tempesta economico-finanziaria di non indifferenti dimensioni. Allora, credo che invece di guardarci alle spalle dovremmo guardare in avanti, capire quali sono i problemi e amo tentare di

di Roma: è stata data la possibilità al Comune di Roma di derogare rispetto al patto di stabilità. Il patto di stabilità è un oggetto misterioso,

è sempre stato applicato in modo stupido, lo ha detto lo stesso presidente Prodi, e nel nostro Paese in modo ancora più stupido rispetto alla possibilità di tentare di premiare realmente gli enti virtuosi rispetto agli spreconi. spreconi. In questa situazione, con la vostra scelta per Roma, intanto avete fatto diventare famoso questo termine e diventa per noi molto più semplice spiegarlo ai cittadini. È incomprensibile immaginare un Paese dove, per rispettare il patto di stabilità, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni non pagano i fornitori. La collega Leddi e anche altri colleghi facevano riferimento al ritardo nei pagamenti. Ebbene, la pubblica amministrazione è in una situazione di difficoltà economica da anni - non sto parlando di questi ultimi mesi - e paga in ritardo.

Se volete tagliare la spesa pubblica bisogna pagare i fornitori, bisogna pensare ad un patto di stabilità che dia questo tipo di risposta. Alcune proposte emendative sono state fatte. So perfettamente che non verranno accolte. So anche, però, che ci sono altri provvedimenti che arriveranno dopo questo decreto e penso che quella sarà l'occasione perché, in modo serio

e che, viceversa, premi gli enti che sono stati virtuosi, che hanno risparmiato e che sono riusciti in questi anni a fare buona amministrazione. Infatti, per assurdo, in questi anni, i meccanismi messi in atto sono stati tali per cui

speriamo veramente che questa situazione di crisi venga affrontata con l'idea di cambiare questo Paese: se è così, noi ci siamo. Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, come ha ricordato nel suo intervento la senatrice Bonfrisco, nel testo originario del decreto anticrisi presentato dal Governo erano stati azzerati i cosiddetti ecoincentivi, cioè gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie che comportano vantaggi dal punto di vista dell'efficienza energetica. Come si sa, alla Camera gli ecoincentivi sono stati reintrodotti, più o meno nella forma originaria. Il Partito Democratico si è battuto con forza per questo risultato, insieme alle principali forze sociali e produttive e a moltissimi cittadini che, in questi mesi, hanno utilizzato

Gli ecoincentivi sono tornati, ma credo che questa vicenda resti sintomatica del modo arretrato ed anacronistico con il quale questo Governo e questa maggioranza guardano al rapporto tra economia ed ambiente, nonché al ruolo delle politiche ambientali in una congiuntura economica difficilissima come quella attuale. Nel corso del 2008 molti italiani hanno utilizzato gli ecoincentivi, facendo un favore a se stessi e un favore al Paese. Peraltro, anche l'argomento per cui i costi delle detrazioni sarebbero un aggravio troppo pesante per le finanze pubbliche, è parzialmente infondato: dei 1.800 milioni di euro portati in detrazione per spese sostenute fra il 2007 e il 2008 - dunque utilizzando gli ecoincentivi introdotti dal Governo Prodi - molti non sono stati sottratti alle entrate dello Stato, per la semplice ragione che senza ecoincentivi una buona fetta di quegli importi non sarebbe stata spesa o sarebbe stata spesa in nero. L'efficienza energetica è uno dei terreni su cui l'Italia ha camminato più lentamente nel confronto con il resto dell'Europa. Eravamo un Paese virtuoso; oggi siamo sotto la media dell'Europa a 15, vale a dire più avanzati dell'Unione europea. Favorire il miglioramento dell'efficienza energetica vuol dire ridurre i costi energetici a carico delle famiglie, ridurre il fabbisogno energetico, migliorare la competitività delle imprese: vuol dire dunque lavorare, al tempo stesso, per migliorare l'ambiente e per rafforzare e modernizzare l'economia. In tutto il mondo occidentale, da Obama - lo abbiamo sentito e letto - a Sarkozy, l'azione di contrasto degli effetti della crisi economica vede proprio l'impegno sul fronte dell'efficienza energetica come uno dei più rilevanti, secondo una ricetta che mescola Keynes con la sostenibilità. In Italia finora non è stato così. Prima col tentativo fortunatamente sventato di boicottare il pacchetto clima, poi con quest'altro infortunio - anch'esso rientrato - che ha visto il tentativo di azzeramento degli ecoincentivi, il Governo ha mostrato una preoccupante e ricorrente abitudine a considerare l'ambiente nemico dell'economia, specie in una congiuntura difficilissima come quella attuale. A chi richiama l'esempio dei piani anticrisi ben altrimenti incisivi e ben diversamente orientati, varati in queste settimane nei principali Paesi industrializzati, dal Governo e dalla maggioranza si risponde, in genere, che l'Italia ha un deficit e un debito pubblico tali da impedire analoghi impegni di risorse. Questo è certamente vero, ma proprio la maggiore fragilità dei nostri conti pubblici dovrebbe suggerire - come ripetutamente ha sollecitato il Partito Democratico, anche con molte proposte specifiche e puntuali di evitare esborsi impropri o tutt'altro che urgenti (penso ad esempio alla cancellazione dell'ICI sulla prima casa per i redditi medio-alti, o alla vicenda Alitalia), e concentrare invece le risorse disponibili nei settori veramente strategici, dove l'effetto anticongiunturale si accompagna ad un effetto di modernizzazione di più lungo respiro. Si tratta dei settori collegati all'ambiente, all'istruzione e alla formazione, alla scienza e alla ricerca, cioè quei settori, disgraziatamente, più penalizzati o più trascurati in questi nove mesi di Governo della destra. La nostra speranza e il nostro appello è che la maggioranza sappia rapidamente correggere questo errore, che forse è mentale prima che politico, e che comporta un grande rischio, cioè che quando la crisi sarà finita

si esce prima e meglio se lo sforzo straordinario, necessario a sorreggere i consumi, la domanda, le imprese, è finalizzato a rendere più efficiente e moderno il nostro Paese. E l'ambiente, e quello che da più parti viene invocato come un *New Deal* ecologico, sono a nostro avviso assi irrinunciabili di questo impegno.

In questa legislatura, dovendo affrontare la crisi, a mio parere il Governo ha saggiamente preso delle decisioni quest'estate, ad esempio anticipando la manovra finanziaria che, per la verità, era molto semplificata,

chiedersi cosa deve fare un Paese privo di risorse pubbliche per recuperare il *gap* infrastrutturale e far ripartire le opere pubbliche necessarie perché costituiscono un volano straordinariamente

stiamo faticosamente cercando di affermare il senso di una rivoluzione culturale, un cambiamento di sistema, di cultura, di approccio attorno a queste problematiche. Nel 2001, signora Presidente,

dovuta alla falsa rivoluzione di Tangentopoli, che aveva creato un clima di terrore nel Paese, alla mancanza di risorse pubbliche o alla macchinosità delle leggi.

aveva fatto sapere che aveva la pistola puntata e stava bene attenta a cosa faceva il Parlamento in quel passaggio importante. Proprio la legge Merloni è all'origine della crisi del sistema infrastrutturale italiano e ha generato la paralisi delle opere pubbliche nel nostro Paese. Dal 2001 al 2006 faticosamente abbiamo cercato di smontare questa legge. Quando si parla di legge obiettivo si fa sempre una semplificazione, perché in realtà il Parlamento in quei cinque anni approvò tre leggi la legge obiettivo, che è una legge delega, il decreto delegato della legge obiettivo e la riforma della legge Merloni, che introdusse per la prima volta un elemento di grande qualificazione,

si sono costruite opere pubbliche con l'approvazione di 2.372 progetti, che hanno dato vita a investimenti di risorse private per 25 miliardi di euro

in termini politici, sono stati anni di paralisi dovuti al protagonismo del ministro Di Pietro, che ha cominciato a cancellare i contratti delle concessionarie autostradali (contratti liberamente sottoscritti dalle parti), compiendo atti illeciti che l'Unione europea ha censurato e comunque pretendendo di comandare il mercato italiano attraverso decreti che intendevano demolire quanto avevamo fatto in precedenza. Dopo la parentesi Di Pietro-Prodi, siamo tornati a conquistare la maggioranza: cosa abbiamo fatto prima di questo decreto? E cosa c'è d'importante in questo decreto, che il dibattito finora non ha evidenziato?

possono proporre agli enti pubblici (e allo Stato nelle sue articolazioni: Comune, Provincia, Regione, ANAS o Ferrovie) opere che neanche sono nel piano programmatico deliberatamente da loro sottoscritto o proposto.

Signora Presidente, lei è stata tanti anni in Europa, quindi forse saprà che siamo l'unico Paese in Europa che dispone di un codice dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, frutto dell'azzeramento di ben 65 leggi preesistenti, che si sommavano proprio nel settore dei lavori pubblici, delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture. Quindi, abbiamo fatto chiarezza normativa, semplificando le norme, e ci accingiamo a

in maniera assolutamente illecita ed illegale, il Ministro della compagine Prodi aveva azzerato tutte le convenzioni in essere nel nostro Paese, liberamente sottoscritte dallo Stato e dalle società concessionarie. Vi è poi la questione

c'è una cosa straordinaria e ormai, visto che domani diventerà legge, possiamo ben dirlo: c'è la possibilità di utilizzare un potenziale enorme, perché il patrimonio della Cassa depositi e prestiti ammonta a 100 miliardi, anche a fini privatistici, nel senso che i privati possono attingere da questo istituto

negli uffici postali, per avere un senso di questo patrimonio. Sapete cosa ha risposto il direttore generale? Sapete quanti sono i libretti a risparmio che affluiscono alla Cassa depositi e prestiti? Signora Presidente, in Italia ci sono 29 milioni di risparmiatori che hanno portato i loro risparmi agli uffici delle Poste *(**Commenti intelligentemente gestiti e saranno gestiti molto bene anche nel futuro, creando che cosa? Creando la BEI italiana. Se faremo le cose ben fatte, avremo a disposizione un istituto di credito che ha il potenziale della BEI; quindi non dovremo più andare a Bruxelles, perché la stiamo facendo in casa. In funzione di cosa? Al fine di creare le condizioni per lo sviluppo economico mirato soprattutto a recuperare questo maledetto *gap* infrastrutturale che abbiamo, che ci siamo creati perché non abbiamo saputo decidere, perché abbiamo premiato la trasparenza sull'efficienza e perché non abbiamo preso nei momenti giusti le necessarie decisioni. Con il decreto-legge in esame, a parer mio, facciamo un altro passo nella giusta direzione.

è già tutto scritto sul risultato finale in Aula del provvedimento in esame. Già sette giorni fa un autorevole quotidiano titolava: «Corsa contro il tempo». Il testo anticrisi appare blindato anche a causa degli strettissimi tempi a disposizione, ma con tutta probabilità il Governo, per risolvere la questione degli errori nel testo licenziato - perché ci sono anche questi ricorrerà ad un provvedimento apposito o ad emendamenti al decreto mille proroghe. Questa è la fotografia del testo di legge oggi in Aula. Così la manovra finanziaria che è stata messa in campo l'estate scorsa e presentata come un'innovazione della sessione di bilancio in termini di anticipazione e di programmazione triennale dimostra oggi tutti i suoi limiti, perché delle due cose l'una: o il Governo a giugno non aveva intuito la gravità della crisi economica di cui pure si intravedevano le forti avvisaglie e non si era preparato a parlarne i colpi, il che di per sé sarebbe già grave; oppure lo sperpero di denaro pubblico che ha segnato le prime scelte di questo Governo appare ancora più irresponsabile. siamo passati dalle leggi finanziarie onnicomprensive del passato ad una manovra economica inconcludente, che continua e si trascina da nove mesi: decreto-legge n. 93, decreto-legge n. 118, legge finanziaria, decreto antibanche. È un fatto certamente grave non solo per la trasparenza e l'approfondimento del processo di formazione del bilancio dello Stato, ma è un fatto ancora più grave, anzi gravissimo, perché in un momento di crisi drammatica il Governo rinuncia ad avere oggi, e a proporre fin da oggi, uno straccio di politica economica capace non dico di risolvere, ma almeno di affrontare una disparità vergognosa che si sta sempre più determinando nelle condizioni sociali ed economiche della nostra gente e del nostro Paese. Al di là dei libretti di risparmio, una famiglia su cinque non può permettersi di acquistare medicine, una su due non riesce a sostenere una spesa imprevista di 700 euro e sette su cento hanno difficoltà a comprare da mangiare. Sono dati ufficiali dell'ISTAT e nei prossimi mesi non è difficile prevedere un quadro ancora più devastante. La recessione è più dura del previsto, il PIL va giù del due per cento, la produzione industriale scende del 13 per cento, le imprese chiudono, la gente perde il lavoro. Sono queste stime della Confindustria, stime che parlano di almeno 600.000 disoccupati in più a breve periodo. E qual è la risposta del Governo? Un ottimismo di facciata, di maniera, incapace di fornire una prospettiva coerente di medio termine. La crisi c'è ma non riguarda solo noi, ci ha ricordato il presidente Berlusconi. Bene, vogliamo guardare agli altri? Berlino ha già varato misure per 32 miliardi, Parigi un piano da 20 miliardi, Londra ha imboccato una strada ancora più impegnativa annunciando il taglio dell'IVA dal 17,5 al 15 per cento. Con il decreto-legge oggi in esame, a mio giudizio, c'è un passaggio preoccupante e discriminante rispetto ai provvedimenti dei mesi scorsi. Abbiamo superato la fase della propaganda, che andava alla ricerca dei sondaggi, dei colpi di scena, del facile consenso ottenuto con i metodi di *marketing* dei precedenti decreti. L'avere eliminato l'imposta comunale sugli immobili per la fascia medio-alta di reddito e di patrimonio è costato allo Stato oltre tre miliardi ed i Comuni vanno ancora alla ricerca delle risorse perdute. dello scorso anno abbiamo detassato straordinari inesistenti. Quante sono le ore di straordinario che hanno potuto usufruire della detassazione? Sono tendenti allo zero. la beffa della *social card* che ha costretto migliaia di cittadini a mettersi in fila per un atto di elemosina di 40 euro. Dai primi dati risulterebbe che al 31 dicembre sono state consegnate soltanto 520.000 *social card* sul 1.400.000 previsto e annunciato. ancora lo *spot* della *Robin tax*, con il rischio concreto che venga scaricata sui consumatori; non è una mia valutazione, non è un mio giudizio, ma è quanto è contenuto nella relazione annuale della Corte dei conti sulle spese dello Stato. il pericolo di alimentare nuove frodi per l'abbandono di ottime regole di contrasto, dalla limitazione nell'uso di assegni e contanti, alla tracciabilità dei pagamenti legati agli elenchi clienti e fornitori. Questo era quello che era stato fatto nei mesi scorsi. Il decreto-legge n. 185 in esame contiene un passaggio preoccupante e discriminante. Prima si toglieva ai poveri per dare ai ricchi; ora si fa finta di dare qualcosa e non si dà nulla. Nel gergo tecnico-commerciale si parla di pubblicità ingannevole. Sul problema della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie arriva un *bonus* da 200 a 1.000 euro a circa sette milioni e mezzo di famiglie; così è stato annunciato. poiché il *bonus* è una misura straordinaria e quindi verrà erogato una volta sola ed è previsto un solo *bonus* per nucleo familiare a seconda dei redditi dell'intero nucleo e della composizione dello stesso,

quindi, di fatto nessuno potrà usufruire di tale misura. Per contro, non ci si occupa dei mutui a tasso fisso che, al contrario, sono gli unici ad essere in questo momento abbondantemente al di sopra del quattro per cento. Sono stati riempiti i giornali con i riferimenti a questa grande possibilità. Un decreto del ministro Tremonti stabilirà, solo dopo il via libera di Bruxelles, il volume d'affari del contribuente nei cui confronti è applicabile la disposizione e ferma restando la relazione tecnica che prevede che bisognerà stimare gli effetti finanziari. Per cui, ad oggi si ipotizza che si debba fissare la soglia ad un importo pari a 200.000 euro:

Non è stata fornita alcuna seria risposta ai lavoratori autonomi che sono stati esclusi dal sostegno fiscale alle famiglie contenuto nell'articolo 1. Perdono quindi la consistente fetta di attività produttiva sostenuta dagli incentivi fiscali (articolo 29), in cambio gli studi di settore diventano una sorta di ultra *minimum tax* facoltativa; viene completato lo smantellamento delle misure antievasione e viene introdotta una sorta di condono personalizzato permanente.

Si tratta infatti di risorse destinate dal Fondo sociale europeo alle Regioni per il periodo 2007-2013 già in parte impegnate che, comunque, non potranno essere spese tutte subito, reddito per i disoccupati se non nell'ambito dei corsi di formazione: ce lo impone l'Europa e i corsi di formazione non sono a costo zero. Le somme effettivamente disponibili, quindi, non dovrebbero superare i 2-3 miliardi Che dire poi del fatto che, dopo che il Ministro dell'economia aveva fatto quasi una bandiera della sua decisione di evitare per la prima volta al Parlamento italiano il classico assalto alla diligenza sulla legge finanziaria, stati assegnati fondi alla fondazione Bietti di oftalmologia di Roma, poco più di 13 milioni di euro per gli eventi sportivi dell'Expo 2015

in Italia, come in altri Paesi, ha individuato un ulteriore trucco per risolvere i problemi di bilancio del Comune di Roma, in modo da far valere una deroga abbondante al Patto di stabilità interno. Questo è il quadro desolante. Signora Presidente, il compito di assumere l'iniziativa spetta al Governo e noi rispettiamo questa sua prerogativa, ma deve fare però prima i conti con sé stesso iniziando da una seria riflessione sui risultati finora prodotti da questa linea di autosufficienza e di autoreferenzialità. A noi spetterà il compito di preparare un'alternativa e di dare nuova fiducia agli italiani che la stanno perdendo.

fa prevalere un atteggiamento aprioristico di rifiuto. Sappiamo bene che la crisi è importante, delicata e globale

in controtendenza, come dicevo prima, rispetto alle perdite di posti di lavoro e ad una cassa integrazione, una mobilità che è purtroppo sempre più ricorrente. Sotto questo punto di vista, valutiamo con estrema preoccupazione il fatto che

come questo provvedimento contiene norme importanti sul rilancio dell'economia. L'articolo 17, ad esempio, prevede la possibilità del rientro in Italia di ricercatori e docenti con specifici

una vera rivoluzione nel rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese: la detassazione, cioè, di microprogetti di interesse pubblico. Viene quindi messo in atto in maniera forte un provvedimento che spinge sulla sussidiarietà di tipo orizzontale. Sappiamo che sono concetti nuovi. Partiamo dal federalismo che vuole portare vicino ai cittadini

con il centro di potere e di controllo, dobbiamo operare con una sussidiarietà di tipo orizzontale. Questo articolo introduce, sotto questo punto di vista, una novità di assoluto rilievo ed interesse. Ci sono anche

Vi è poi una parte che riguarda il Patto di stabilità speciale con una deroga molto particolare per il Comune di Roma, che ovviamente non va nel senso che vogliamo. Questo sicuramente dovrà essere rivisto e corretto per un equilibrio ed equità rispetto a tutti

il World Economic Forum, il cui tema è importante: ridisegnare il mondo del dopo-crisi. Su questo penso che veramente si stanno muovendo Parlamento e Governo. Con questi provvedimenti abbiamo affrontato

Dal Word Economic Forum e da ciò che stanno predisponendo anche Parlamento e Governo partiranno provvedimenti per il dopo-crisi. Ci stiamo muovendo con senso di responsabilità e i cittadini stanno vedendo e apprezzando il lavoro del Governo e del Parlamento.

vedo che è presente in Aula il ministro Vito, il che mi dice che molto probabilmente questa sera sarà posta la fiducia. Quindi la nostra discussione probabilmente finisce questa sera Ne approfitto solo per dire che molto probabilmente anche in questo caso si sta perdendo un'occasione per un confronto serio e approfondito sulla situazione del Paese. Se diffido degli entusiasti, diffido anche dei catastrofisti allo stesso modo: non mi iscrivo a nessuno dei due partiti. Cercherò però di proporre due o tre ragionamenti, perché mi interessa che

se ognuno di noi può dare un contributo per andare nella direzione giusta, siamo qui, cerchiamo di darlo, cerchiamo di fare la nostra parte e di dare anche dei suggerimenti utili a superare questa situazione di difficoltà. Poiché non sono né un catastrofista né un entusiasta, so benissimo che una crisi come quella che abbiamo dinanzi non si risolve solo in Italia e solo con i provvedimenti che può porre in essere il Governo italiano: è una crisi globale, mondiale,

ma secondo voi questo provvedimento è adatto ad affrontare una crisi che prevede per il 2009 un calo della produzione industriale del 16 per cento? Un calo di due punti del prodotto interno lordo lordo lo affrontiamo con i provvedimenti contenuti in questa manovra? Non lo so, me lo auguro, magari fosse così. Gli entusiasti dipingono

500.000 (e stanno crescendo del 56 per cento) le richieste di cassa integrazione (cresce più quella ordinaria di quella straordinaria).

Costa 4-5 miliardi, però in una situazione come questa ci vuole senso di responsabilità, se non vogliamo dividere il Paese e lo vogliamo tenere unito. Perché per affrontare una crisi così occorre tenere unito il Paese: guai se si dividesse il Paese di fronte ad un crisi del genere. E per tenerlo unito bisogna dare una risposta adeguata a coloro che perderanno il posto di lavoro, a coloro che andranno in cassa integrazione e a tutte quelle famiglie che si troveranno in difficoltà.

a diminuire le tasse ai ceti più deboli, cioè al lavoro dipendente, al lavoro precario; facciamo un'operazione di riduzione delle tasse sui Servono 4-5 miliardi per fare questa operazione. I soldi per gli ammortizzatori sociali e per la riduzione delle tasse sui salari si devono trovare; se un Paese vuole stare unito in una situazione di crisi come questa i soldi per queste cose li deve trovare.

sgravi ai redditi più bassi, alle famiglie e ai redditi che hanno bisogno di avere uno sgravio fiscale per poter alimentare anche i consumi e per poter fare una vita dignitosa in una situazione di crisi come quella che abbiamo davanti. Servono 4-5 miliardi. Passando al tema rifaccio ad una cosa la cui citazione in questo momento fa discutere in positivo e in negativo e rischia di dividere il Paese. La crisi dell'auto

su come affrontare la crisi dell'auto e si stanno discutendo le varie soluzioni dei vari Paesi. Cosa va a proporre l'Italia? Noi saremmo curiosi di saperlo. Quali sono le proposte che l'Italia mette sul piatto della bilancia dell'Europa per dire che noi siamo pronti per affrontare la crisi dell'auto in un certo modo?

contribuire a questa discussione, che è importante. Sarebbe utile, quindi, che attorno a uno dei settori più importanti dell'industria del nostro Paese ci fosse un confronto e un dibattito.

Ieri sera, parlavo con un imprenditore che mi ha detto: sapete qual è problema delle piccole e medie imprese? Che le banche non danno loro i soldi. Che le banche non danno loro i soldi. Diceva che nel settore tessile e nel segmento medio della produzione ha un'azienda in Italia e una in Cina: per fortuna che con quella in Cina

Le banche non gli danno i soldi. Sono questi i problemi concreti del Paese. Vogliamo mettere un po' di risorse fresche perché le piccole e medie imprese possano

Questo voto sarà infatti la dimostrazione di un'assunzione di responsabilità, da parte di quest'Aula e da parte del Parlamento, dopo il voto della Camera, davanti a una crisi rispetto alla quale l'intera classe politica deve agire. in esame intende contrastare una difficile situazione economico-finanziaria agendo su due lati, quello del consumatore e quello delle imprese, tramite una serie di misure che vogliono infondere fiducia fiducia ai due comparti più importanti dell'economia nazionale, aiutando sia chi produce sia le famiglie. Si tratta di

da parte del Governo; è stato introdotto un nuovo modo di concepire i conti dello Stato nella congiuntura che stiamo vivendo, introducendo una manovra di bilancio che non si esaurisce nel giro di pochi mesi, ma una finanziaria permanente che si sviluppa nell'arco di un triennio. Questo è un atteggiamento responsabile ed attento verso gli sviluppi, anche quelli imprevedibili, che possono verificarsi nei prossimi mesi.

che si è rivelata di assoluta importanza rispetto a una crisi internazionale che è venuta dopo, in termini cronologici. Nella strategia tracciata dall'Esecutivo si inserisce questo provvedimento anticrisi, che ha un duplice obiettivo: sostenere la domanda e favorire lo

di settore. Tale revisione costituisce un'anticipazione di quel federalismo fiscale che ha iniziato il suo *iter* in quest'Aula la settimana scorsa, perché gli indici di normalità economica vengono stabiliti tenendo conto del territorio, regionalmente; è infatti evidente che essi non possono essere stabiliti su scala nazionale. Inoltre, è previsto il potenziamento finanziario dei confidi,

per tutti gli imprenditori un tema di vitale importanza. Infine, vorrei menzionare l'IVA per cassa, che non mi sembra una misura da considerare con leggerezza. L'IVA per cassa diventa strumentale, cancellando la sperimentazione dal 2009 al 2011 e consentendo

tra contribuenti e pubblico erario. Non va dimenticata la dichiarata disponibilità del Governo, e del ministro Tremonti in particolare, a sostegno delle piccole e medie imprese, che - lo sappiamo bene tutti in quest'Aula - rappresentano l'ossatura produttiva del nostro Paese. Non sono dimenticate: ci sarà un provvedimento fatto

tante volte auspicato), purché il "rosso", certo, non duri più di trenta giorni perché ci sono dei limiti, evidentemente, in questo momento. Sono nulle anche numerose clausole sfavorevoli ai clienti delle banche, come quella che prevede una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi a prescindere dall'effettivo prelevamento prelevamento dei fondi o quella che prevede una remunerazione alla banca indipendentemente dalla durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, salvo che non ci siano corrispettivi predeterminati con patti scritti non rinnovabili. Queste sono misure evidentemente importanti per il settore delle piccole e medie imprese. Inoltre si è parlato dello sconto del 55 per cento sulle spese di riqualificazione energetica degli edifici, che sono state corrette. E poi c'è tutto il capitolo delle disposizioni dedicate sono state elencate da chi mi ha preceduto. il potenziamento finanziario dei confidi. Per i confidi è stato potenziato il fondo di garanzia con un importo massimo di 450 milioni di euro, mentre la garanzia è stata estesa anche alle imprese artigiane. Si tratta di una norma importante: attraverso il sostegno all'attività di questi organismi si vuole raggiungere l'obiettivo di facilitare e rendere meno oneroso, proprio per le piccole e medie imprese, l'accesso ai finanziamenti bancari. Non dimentichiamo, poi, l'incentivo per il rientro in Italia dei ricercatori che risiedono all'estero: viene previsto che i loro redditi siano fiscalmente imponibili solo

Se ne è parlato, ha sollevato l'argomento il senatore Stradiotto. Non dimenticate che è prevista la cessione *pro soluto* dei crediti verso la pubblica amministrazione, cioè i crediti potranno essere venduti e le aziende potranno immediatamente avere a disposizione che deriva dalla cessione. Non sono state dimenticate neppure le grandi imprese, perché si parla delle modifiche al testo unico della finanza per rendere applicabili le regole relative alla difesa società oggetto di OPA soltanto qualora previste dagli statuti delle società. Anche questo è importante, il Governo ha deciso, attraverso questa misura, di difendere anche le grandi aziende italiane, il cui valore è fortemente sceso a causa della crisi in atto, rendendole quindi appetibili

Il senatore Grillo ci ha detto qual è l'entità dei fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale, che ora possono essere utilizzati anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della Cassa depositi e prestiti nei confronti di Stato,

che mira a ridare fiato ad un settore e ad imprese che devono stare anch'esse sul mercato. Intendo dire che questo provvedimento è ampio; ci sono disposizioni e interventi in tutti i settori. Certo, non possiamo non possiamo risolvere la crisi internazionale in atto con questo decreto; ma dal decreto si ricava una strategia ispirata ai criteri di equilibrio e buona finanza, assolutamente indispensabili per superare questa crisi.

mondo e non possiamo quindi assolutamente essere aperti - e mi ricollego anche alle proposte del senatore Mercatali - ad interventi che aumentino il deficit pubblico. Su questo è chiaro che non potremo mai dialogare.

Com'è noto, Presidente, il provvedimento contiene importanti norme a sostegno delle famiglie e delle imprese per uscire dalla crisi economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese. Il decreto però è praticamente alla vigilia dei termini costituzionali di scadenza per la sua conversione in legge che, com'è noto, cadono il prossimo 28 gennaio.

senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Atto Senato n. 1315), nel testo identico a quello approvato dalla Camera

finestra"). Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge recante norme in funzione anticrisi, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. La discussione generale sulla fiducia si svolgerà tra domani mattina e domani pomeriggio per complessive 3 ore e mezza. Le dichiarazioni di voto di voto avranno luogo nella seduta pomeridiana di domani, a partire dalle ore 18. Seguirà la votazione per appello nominale intorno alle ore 19. In apertura della seduta antimeridiana di domani, che avrà inizio alle ore 10,30, la Presidenza ricorderà il «Giorno della Memoria». Successivamente, potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per dieci minuti ciascuno. Nella seduta antimeridiana di mercoledì 28 gennaio, con inizio alle ore 10, sarà discusso il disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità. per la presentazione degli emendamenti su tale provvedimento è anticipato alle ore 13 di domani. Per il resto, il calendario rimane invariato, salvo l'inserimento nella seduta antimeridiana di giovedì 29 del Documento 6-*ter*, n. 5, in materia di insindacabilità, che sarà esaminato a conclusione della discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sull'elezione contestata nella circoscrizione Estero.

inizio il mio intervento dando una buona notizia al Parlamento. Non sempre ne ho l'occasione. A seguito delle varie interrogazioni parlamentari, mozioni, conferenze stampa, manifestazioni pubbliche che sono state sostenute dalla stragrande maggioranza dei parlamentari italiani, finalmente l'organizzazione dei

hanno avuto e giocato negli ultimi quattro mesi, anche attraverso una delegazione, che mi ha visto presente in prima persona, che si è recata in Iraq al campo di Ashraf. La seconda questione riguarda i nostri lavori della settimana prossima. Capisco che quanto ci è stato comunicato stamani

e più volte l'ho già chiesto - che in occasione del dibattito che si svolgerà in merito alla ratifica di quel Trattato si possa dare quanta più possibilità agli italiani di conoscere ciò che il Governo, in un momento di enorme crisi, ha deciso di fare. Ci viene raccontato che la crisi è iniziata durante l'estate; il Trattato è stato firmato il 30 agosto. Quindi, già si sapeva che le casse dello Stato sarebbero state vuote. Pertanto, far sapere come vengono utilizzati questi soldi, che ammontano a 250 milioni di

che in qualche modo hanno preparato ciò che avviene oggi, cioè il dilagare della crisi industriale e occupazionale a Torino e in Piemonte dovuto specialmente alle questioni che riguardano un altro settore, quello metalmeccanico. Segnalo, dunque, due punti di crisi